Signor Presidente, rappresentanti del Governo, ministro Finocchiaro, colleghi senatori, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea è stato approvato dalla Camera dei deputati il 12 ottobre scorso e trasmesso al Senato il giorno successivo. La Commissione affari costituzionali ne ha iniziato la trattazione il 17 ottobre e ha concluso i suoi lavori nella seduta di ieri, lunedì 23 ottobre. Pur tenendo conto dei tempi serrati di esame, è stata mia cura, in qualità di Presidente, garantire il rispetto delle prerogative dei Gruppi di maggioranza e di opposizione, organizzando i lavori affinché fossero assicurati spazi adeguati a tutte le fasi della sede referente, con particolare riguardo alla discussione generale, senza trascurare le istanze, pervenute dai Gruppi, finalizzate a un approfondimento dei contenuti del testo approvato dalla Camera, attraverso l'audizione di costituzionalisti. Anche la fase di esame e di votazione degli emendamenti si è svolta in tempi che considero congrui. Nel riferire sul disegno di legge n. 2941, desidero però compiere alcune considerazioni di carattere generale. È a tutti noto che i vigenti sistemi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si basano sulle normative risultanti dagli effetti di annullamento prodotti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. All'esito di queste pronunce, le leggi elettorali per i due rami del Parlamento presentano differenze significative, suscettibili di produrre risultati eterogenei. Potrebbero dunque determinarsi effetti incongrui rispetto all'assetto delle future Camere, con possibili conseguenze negative sulla stabilità e sull'efficienza del sistema istituzionale. Il Presidente della Repubblica ha manifestato in più occasioni le sue preoccupazioni al riguardo, invitando il Parlamento, nel rispetto delle prerogative proprie del potere legislativo, affinché sia compiuto ogni sforzo per approvare normative tra loro coerenti. In questo scorcio di legislatura, il Parlamento è chiamato a un gesto di responsabilità istituzionale, intervenendo per superare le più marcate criticità della vigente legislazione elettorale. Sono consapevole che, nell'ambito della riflessione scientifica su questo tema, si registra una convergenza circa l'esigenza che le regole elettorali siano quanto più possibile stabili e che, in ogni caso, siano modificate in una fase temporalmente distante da quella nella quale dovranno essere applicate. Pur tuttavia, occorre considerare che questo assunto, certamente condivisibile in via generale, cede di fronte ai tratti particolari e anomali del contesto attuale, soprattutto in ragione, come ho detto, dell'eterogeneità dei due sistemi elettorali, tanto più evidente ove si consideri che, dopo l'esito del *referendum* del 4 dicembre scorso, le due Camere conservano lo stesso potere ed esercitano le medesime funzioni. In particolare, sono entrambe titolari del potere di accordare e revocare la fiducia al Governo è proprio in considerazione di tale fondamentale prerogativa costituzionale che le differenze tra i due sistemi risaltano con estrema evidenza. Le più significative differenze tra i due sistemi elettorali attualmente vigenti sono le seguenti. Al Senato sono ammesse le coalizioni tra liste, mentre alla Camera dei deputati non sono consentite. Per l'elezione del Senato trova applicazione un articolato sistema di soglie di sbarramento, mentre per l'elezione della Camera dei deputati è previsto che possano accedere alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, con eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, per le quali vige un sistema *ad hoc*. Per quanto riguarda le preferenze, per l'elezione del Senato, all'esito della sentenza n. 1 del 2014 è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993, come modificato dalla legge n. 270 del 2005, nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere la preferenza per i candidati. Per l'elezione della Camera dei deputati, invece, la legge n. 52 del 21 dicembre 2015 prevede che ogni lista sia composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, in favore dei quali l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza. prevede norme a garanzia della rappresentanza di genere, mentre nella legge elettorale per l'elezione del Senato non è prevista alcuna disposizione di tale tenore. Infine, per l'elezione del Senato non è prevista l'attribuzione di alcun premio di maggioranza, mentre per l'elezione della Camera dei deputati persiste un premio di maggioranza, seppure solo eventuale, in favore della lista che abbia raggiunto, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei Dalla descrizione delle differenze tra i sistemi elettorali per l'elezione dei due rami del Parlamento emerge, con evidenza, l'urgenza di un intervento. Credo, quindi, che debba essere raccolto l'invito del Capo dello Stato. Come ho già detto, il Parlamento è chiamato a un atto di responsabilità, approntando, nei limiti di tempo che ha a disposizione e tenendo conto del quadro politico attuale, una legislazione elettorale compiuta e coerente. Certamente le soluzioni potevano essere le più varie: formule elettorali maggioritarie fondate su collegi uninominali; formule elettorali proporzionali, al cui interno si apre un ampio spettro di possibili varianti; formule miste. Purtroppo, il tempo che residua prima della fine naturale della legislatura non consente ulteriori indagini sulla scelta migliore. Occorre, invece, in questa fase della legislatura, mettere in sicurezza il sistema, adottando una normativa coerente, quanto più possibile condivisa e in linea con le indicazioni generali che emergono dalla lettura delle sentenze della Corte costituzionale in materia. Alla luce di questi canoni, credo che il testo ora all'esame del Senato rappresenti un punto di equilibrio. Qualora il disegno di legge sia approvato, avremmo sistemi elettorali uniformi per i due rami del Parlamento. Come emerge dalla lettura dei lavori parlamentari presso la Camera dei deputati e come è stato confermato dall'andamento dei lavori in Senato, è maturata su questo testo una positiva convergenza tra forze di maggioranza e alcune forze di opposizione. Sono rispettati alcuni dei più significativi principi desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale, con particolare riguardo al principio della rappresentanza e al principio di conoscibilità del candidato da parte dell'elettore. Riferisco dunque, nel dettaglio, sul provvedimento in esame. Il disegno di legge delinea un sistema elettorale misto: l'assegnazione di 232 seggi alla Camera dei deputati (comprensivi di un collegio in Valle d'Aosta e di 6 collegi in Trentino-Alto Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di un collegio in Valle d'Aosta e di 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato: l'assegnazione dei restanti seggi avviene nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento. Sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. dei deputati, ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali e in uno o più collegi plurinominali. I collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. La determinazione dei collegi uninominali, così come quella dei collegi plurinominali, è rimessa a una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali, costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. Nella disposizione di delega al Governo, viene precisato che la determinazione dei collegi plurinominali avviene in modo che «tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio». Il numero dei collegi uninominali è dunque determinato dalla legge, mentre il numero dei collegi plurinominali, risultanti dall'aggregazione di uno o più collegi uninominali, è rimesso al decreto legislativo di cui all'articolo 3, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi previsti. Al Senato il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni, corrispondenti al territorio di ciascuna Regione. Ciascuna circoscrizione regionale è suddivisa in collegi uninominali e in uno o più collegi plurinominali. I collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; la determinazione dei collegi uninominali - così come quella dei collegi plurinominali - è rimessa, come per la Camera dei deputati, a una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Anche al Senato i collegi plurinominali sono costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a I criteri e principi direttivi per l'attuazione della delega sono in gran parte i medesimi di quelli previsti per la determinazione dei collegi della Camera. Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intenda presentarsi alle elezioni, sia alla Camera, sia al Senato, è tenuto a depositare il proprio contrassegno e a indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno nei termini previsti; contestualmente al deposito del contrassegno, deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica. Sia alla Camera sia al Senato i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali. Sia alla Camera sia al Senato, in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, indipendentemente dal numero di seggi assegnato il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a due né superiore a quattro. In sede di presentazione della lista sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale; ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione. La lista, sia alla Camera sia al Senato, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nei medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico Comune, iscritti nelle sezioni elettorali di quel collegio plurinominale. Il testo reca inoltre una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per definire le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste. Nel caso di liste collegate in coalizione, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali, ad eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, che possono presentare separatamente il proprio candidato. Sia alla Camera sia al Senato nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di cinque. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale. Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere. In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere. Al contempo, alla Camera è previsto che, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni. Al Senato le medesime previsioni sono stabilite a livello regionale e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime. Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati - da due a quattro - nel collegio plurinominale. Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. Sono previste, altresì, nuove disposizioni che attengono alla base dello spoglio delle schede e del relativo scrutinio. In particolare, è previsto che le schede elettorali siano provviste di un tagliando antifrode con codice progressivo alfanumerico. Come già ricordato, nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più giovane per età. Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali, alla Camera il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Le soglie di sbarramento sono del 3 per cento a livello nazionale per le liste singole e del 10 per cento a livello nazionale per le coalizioni (purché almeno una lista intracoalizione raggiunga il 3 per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell'uno per cento. Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche: il requisito previsto è in tal caso il raggiungimento del 20 per cento a livello regionale o aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali. Al Senato l'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata con metodo proporzionale e avviene a livello regionale. Accedono al riparto le coalizioni di liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e le liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella Regione o, per le minoranze linguistiche, aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali. Al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. Sono altresì specificate le modalità con cui si procede, sia alla Camera sia al Senato, alla proclamazione degli eletti in caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale. Subentrano dapprima i candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione. Esaurite tutte le liste della circoscrizione, subentrano i cosiddetti "migliori perdenti" (sulla base della graduatoria redatta dall'ufficio elettorale circoscrizionale) nei collegi uninominali del collegio plurinominale e, successivamente, i migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione. Si procede poi proclamando eletti i candidati presentati dalla lista nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni. In caso di ulteriore incapienza, si procede proclamando eletti i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinominale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione. Nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, subentrano i migliori perdenti nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni e, infine, i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni. Per il Senato, si procede analogamente, con la differenza che non si applicano le norme che consentono il subentro di candidati di altre Regioni. Riguardo alla disciplina dei cosiddetti subentri nel caso in cui un seggio rimanga vacante, anche per causa sopravvenuta - si prevede che il seggio sia attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione. un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive. L'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 contiene disposizioni transitorie. Alcune di tali disposizioni riguardano le sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature nelle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge. In particolare, viene modificata la disposizione recata dal comma 36 della legge n. 52 del 2015, in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, prevedendo che tale esonero si applichi per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, per la Camera e per il Senato, ai partiti o ai gruppi politici costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data del 15 aprile 2017. per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione alla Camera dei deputati (almeno 1.500 e non più di 2.000 sottoscrizioni degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio plurinominale) sia in ogni caso ridotto alla metà. Una norma in parte analoga è prevista per il Senato, dove è stabilito che il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature (le stesse fissate per la Camera, quindi da 1.500 a 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio plurinominale) è ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni. Il comma 7, invece, riguarda i soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste: esclusivamente per le prossime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge sono abilitati, oltre ai soggetti già previsti, anche gli avvocati abilitati al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto della circoscrizione elettorale. Quanto ai soggetti abilitati, il testo aggiunge - a regime - i sindaci metropolitani e i componenti della conferenza metropolitana, nonché i consiglieri metropolitani, alla luce dell'istituzione delle Città metropolitane operata dalla legge n. 56 del 2014. Sono, inoltre, previsti i tempi per l'esercizio del diritto di opzione per il voto degli italiani temporaneamente all'estero. Altre norme intervengono, invece, sui requisiti di elettorato passivo per la circoscrizione Estero. In primo luogo, non è più richiesto il requisito della residenza nella ripartizione della circoscrizione Estero per chi intende candidarsi. Al contempo, si prevede che gli elettori residenti in Italia possano essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero. Gli elettori residenti all'estero possono, a loro volta, essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero (non è modificato l'articolo 8, comma 4, della legge n. 459 del 2001 che prevede che gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione per esercitare il diritto di voto in Italia, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale). Infine, si prevede che non possano essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto, nei cinque anni precedenti la data delle elezioni, cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un Paese della circoscrizione Estero. È prevista, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Come ho già detto, la circostanza che la legge elettorale sia approvata dal Parlamento a pochi mesi dalla scadenza naturale della legislatura si giustifica per la particolarità dell'attuale contesto politico istituzionale. Peraltro, come segnalato nel corso delle audizioni da alcuni costituzionalisti, la modifica dei sistemi elettorali - contrariamente a quello che si pensa o si teme - quasi mai favorisce i fautori della riforma, dal momento che tra sistema elettorale e sistema politico sussiste un rapporto circolare di reciproca influenza. Il sistema politico si modella sulla base della legge elettorale adottata, modificando l'offerta politica in forme che non sono conoscibili *ex ante*. Ritengo pertanto necessario che si sgombri il terreno da questa insidiosa speculazione politica, smentita, nella sua veridicità, dalle vicende costituzionali italiane degli ultimi Al contrario, ritengo - al di là delle legittime posizioni assunte dai diversi Gruppi parlamentari - che sia in ogni caso meritevole di considerazione il fatto che il Parlamento abbia assunto la responsabilità di legiferare in materia elettorale, adempiendo con scrupolo ad un dovere costituzionale che ne riqualifica ruolo e azione. Il tentativo di dotare le Camere di leggi elettorali più adeguate e coerenti risponde anche a un'esigenza di respiro costituzionale, ovvero che le leggi elettorali siano di estrazione strettamente parlamentare, non essendo opportuno - come peraltro sottolineato in diverse sedi - che le regole fondamentali dell'agire politico, segnatamente quelle che definiscono le modalità di formazione degli organi elettivi, siano prodotte in sedi diverse dal Parlamento. *(Applausi

«Fare una legge in Parlamento, in questo momento, in questo momento storico, che va contro il Movimento 5 Stelle è una cosa pazzesca, criminale, una sciocchezza. Me la potrei cavare così, ma io dico che è anche immorale. Non si fa una legge sei mesi prima delle elezioni per punire il Partito». « (…) sono strabiliato del fatto che tutti accettino che alla vigilia delle elezioni si fa una legge che va in tasca al partito che potrebbe essere quello di maggioranza relativa. Con che faccia, partiti che ricevono un premio in seggi che li sovrarappresenta rispetto a un eventuale partito di maggioranza relativa, poi si mettono a costruire un Governo?». A parlare così non è un feroce avversario della maggioranza, ma un commentatore amico di questo Governo, come l'ex direttore de «Il Corriere della Sera», Paolo Mieli. Il crimine comporta dolo, cioè volontà, una volontà porca, «una porcata», appunto, come Calderoli definì lo stravolgimento della sua legge elettorale nel 2005. Questo non gli impedì di votarla, così come oggi la Lega sta avallando questa nuova porcata. È naturale, direi genetico:

Se vi ripugna il parallelismo, posso tornare a chiamarvi criminali. Quando, dopo le tre votazioni con il Porcellum, la Corte costituzionale lo dichiarò incostituzionale, chiedemmo di tornare immediatamente al voto con la legge che la Consulta finalmente aveva restituito al Paese. Lo affermò qui in Senato, in audizione, anche il professor Pace. Invece, i figli del Porcellum che hanno tentato di divorarsi la Costituzione, hanno escreto una nuova legge incostituzionale: l'Italicum. Quando, poi, nuovamente, la Corte lo ha cassato, restituendoci un modello elettorale tuttora vigente e immediatamente applicabile, rappresentativo della volontà popolare e funzionale a dare governabilità - magari al Movimento 5 Stelle non lo hanno più voluto e stanno intentando una terza porcata: il Porcellum-Rosatellum. Lo fanno a pochi mesi dal voto, con il ricatto del voto di fiducia che il Governo ha posto per ben tre volte alla Camera. Ieri ci siamo sentiti dire dal Governo che è intervenuto solo perché richiesto dalla Camera dei deputati: bugia! Lo ha chiesto il Partito Democratico. Qui al Senato il Governo lo ha annunciato in anticipo, senza che alcuno lo avesse invocato, tradendo la sua frenesia, come ho detto ieri Perché è grave l'apposizione del voto di fiducia? Perché l'articolo 72 della Costituzione per le leggi elettorali obbliga ad adottare la procedura normale di esame e di approvazione diretta, senza l'intervento del Governo a ricattare il libero convincimento dei parlamentari. Lo chiarì già nel 1980 l'allora presidente Nilde Iotti: nei Regolamenti parlamentari la fiducia non era nella seconda parte del Regolamento, dedicata al procedimento legislativo. È un fatto particolare, a parte. hanno fatto peggio: la fiducia è stata imposta su una legge mai discussa in Commissione, senza audizioni né simulazione dei suoi effetti. Con la fiducia non si sono potuti votare emendamenti fondamentali per restituire a questo scellerato testo una decenza costituzionale. Anche qui al Senato la discussione generale in Commissione è avvenuta in un clima surreale, nella totale assenza di tutti i membri della maggioranza, che ha annunciato poi che avrebbe respinto in fase emendativa ogni proposta,

l'apposizione del voto fiducia; con la fiducia il Governo se ne fotte dei tempi di lavoro in Commissione; se ne fotte delle prerogative del Parlamento e, soprattutto, dei milioni di italiani stremati dalla crisi e annichiliti dalle ricette economiche di questi cinque anni, che vedono in questi giochetti l'ennesimo arrocco del Palazzo e un sistema, quello che voi rappresentate, ormai alla canna del gas.

il voto congiunto senza scorporo viola il principio di eguaglianza, sancito dagli articoli 3 e 48 della Costituzione; i voti degli elettori di un candidato nominale vincente, nonostante abbiano già trovato rappresentanza, vengono nuovamente conteggiati per la quota proporzionale.

Il sistema di trasposizione dei seggi dai livelli superiori ai collegi plurinominali e le sue conseguenze in tema di ammissibilità delle liste boccate viola il principio espresso dalla Corte costituzionale in materia di conoscibilità degli effetti del voto.

Ciò significa che faranno la fisarmonica, stringeranno, allargheranno, cuciranno i collegi per determinare esattamente l'elezione dei loro nominati, facendo sì che siano votate in Parlamento le persone che domani saranno pronte ad alzare la mano a bacchetta. In questa operazione si avvarranno di una commissione di esperti nominata dal Governo, e quindi non neutrale, come abbiamo visto in passato. Le soglie nazionali al Senato contrastano con l'articolo 57 della Costituzione che fa riferimento alla base regionale. Chiedo a voi, colleghi, se siete disposti, quand'anche foste rieletti, a rientrare in queste Aule

Lo abbiamo visto in Commissione con la discussione surreale nel vuoto totale, tanto che abbiamo detto al Presidente che ce ne andavamo perché non vi era ascolto, non vi era la minima decenza, ma solo il vuoto. Lo abbiamo visto con gli emendamenti respinti a prescindere, con il Governo che si proclama neutrale e invece poi pone la fiducia. Abbiamo chiesto al Capo dello Stato di esercitare una *moral suasion*, prima ancora del suo potere di rinviare alle Camere. Oggi, infatti, si può evitare una vergogna: siamo noi responsabili di fermare o perpetrare l'umiliazione dei cittadini, che già tre volte sono stati umiliati e portati a votare con il Porcellum, che sono stati umiliati dall'ennesima legge burla - l'Italicum - valida solo per una Camera, e dalla riforma di un terzo della Costituzione, portata avanti a colpi di maggioranza,

in quattro anni e mezzo: uno ogni tre giorni. E adesso umiliate ancora gli italiani con l'ennesima legge che porterà un Parlamento di nominati,

Dunque, perché non si alza il capogruppo Zanda e non dice che l'accordo, raggiunto con Berlusconi, Alfano e Salvini (e mettiamoci pure dentro Verdini), è servito, perché è questo ciò che vogliamo: un Parlamento ancora più servo!

di farsi dichiarare incostituzionale per la terza volta una legge elettorale. Ciò che è accaduto nel nostro Paese, ovvero la dichiarazione di

il candidato del collegio uninominale eletto con il sistema maggioritario oppure una lista di partito o movimento politico in collego plurinominale, i cui candidati risulteranno eletti con metodo proporzionale. L'elettore può optare per un candidato nel collegio uninominale, e quindi votare automaticamente anche per tutte le liste ad esso collegate, oppure ne indicherà una, quindi un collegio uninominale

ci sarà immediatamente uno slittamento automatico della volontà dell'elettore da un determinato candidato del collegio uninominale a liste non votate dall'elettore stesso, bensì in proporzione ai voti attribuiti.

il proprio voto utilizzato per far eleggere persone che la pensano all'opposto e che magari hanno combattuto per tutta la vita.

evitare la disuguaglianza del voto e per fare in modo che il voto possa essere libero. Per cui posso votare un determinato candidato nel collegio uninominale perché quella persona mi convince, ma magari voglio esprimere il mio voto liberamente per un'altra lista. Ma questo non sarà possibile,

eletto produrrà, in quale Regione o circoscrizione. Questo è l'altro meccanismo assurdo che ci troviamo di fronte. Arriviamo poi alla chicca finale sul Trentino-Alto Adige.

tra collegio nominale e collegio plurinominale e quello eletto proporzionalmente. Signor Presidente, gli elementi sono moltissimi e arrivo a un altro fatto. questioni pregiudiziali, ma dei fatti sono già avvenuti: alla Camera si è seguita la procedura ordinaria per approvare la legge elettorale? Assolutamente no.

abbiamo cominciato a illustrare il primo emendamento, il Governo - che poi ha detto che non c'entrava nulla - aveva già dichiarato fuori, inventandosi un numero esorbitante di voti segreti, che già si predisponeva al voto di fiducia. È questa la procedura ordinaria cui la nostra Costituzione chiede di attenersi per approvare la legge elettorale? È per questo motivo che il

di questo ennesimo schiaffo alla Costituzione - quali saranno i costi che pagherete. Poi c'è una maledizione sulle leggi elettorali.

su un aspetto assolutamente essenziale che è quello legato alle soglie di sbarramento. Noi ci troviamo - com'è già stato ricordato dalla collega De Petris - in un sistema misto. misto. I sistemi elettorali, o meglio, le formule elettorali si dividono da sempre in due grandi famiglie: la famiglia delle formule maggioritarie e quella delle formule proporzionali. È vero che dagli anni del secolo scorso tutte le innovazioni in tema di leggi elettorali nel mondo sono state tese a superare i modelli originali, solamente maggioritario o solamente proporzionale, per creare le famiglie dei sistemi misti

non sono un correttivo maggioritario, ma un correttivo al sistema proporzionale per raggiungere l'obiettivo di di ridurre la frammentazione partitica e, quindi, dei Gruppi parlamentari. L'obiettivo dei sistemi proporzionali è fotografare l'opinione prevalente del corpo elettorale e restituire una fotografia più aderente possibile alla realtà che è fuori dalle Aule del Parlamento. L'intervento in riduzione della frammentazione avviene con

una truffa semantica nei confronti dell'elettore che comincia proprio dalle coalizioni che richiamano il sistema del Mattarellum, ma nel Mattarellum le coalizioni avevano il simbolo di coalizione: la scheda alla Camera con il simbolo della coalizione e la scheda al Senato con il simbolo della coalizione. caso avremo coalizioni non coalizioni, senza simbolo, senza programma comune e senza *leader* designato. simili - e rubo un'immagine usata dal collega Migliavacca in Commissione - a liste apparentate che non a liste in coalizione. Ebbene, nonostante il carattere destrutturato delle coalizioni, i voti ottenuti

del quale «il voto è personale ed eguale, libero e segreto». Da questo punto di vista, falsificazione e manipolazione rappresentano una distorsione che ci porta a chiedere all'Assemblea di non procedere all'esame dell'atto Senato n. 2941.

per la seconda volta ci troviamo davanti all'esame di un disegno di legge elettorale. Nella prima occasione, in dissenso da quello che era allora il mio Gruppo di appartenenza, mi sono opposta come ho potuto - ci siamo opposti come abbiamo potuto - ai cosiddetti emendamenti premissivi,

che da più parte viene denunciato. Normalmente la Corte costituzionale si pronuncia su aspetti che vengono sottoposti in maniera puntuale, ma in realtà è il sistema che deve rispondere alla normativa e ai principi costituzionali. Un'altra considerazione emersa è che gli effetti che si determinano in concreto, con i risultati elettorali, incidono sulla valutazione complessiva della ragionevolezza di un sistema. E qui abbiamo un sistema maggioritario, ma soprattutto, in maggior parte, un sistema proporzionale; scommessa e la nostra valutazione è che esso potrebbe non garantire né la rappresentatività, né la stabilità del Governo, con un sacrificio degli altri beni giuridici che risultano ristretti, che risulterà non rispondente alla necessità o all'opportunità di contemperare rappresentatività e governabilità. Rispetto alle stesse procedure utilizzate per l'approvazione, in particolare l'apposizione della fiducia in una materia strettamente parlamentare - lo dico davanti al Ministro dei rapporti

un contrasto con l'articolo 72, ultimo comma, della legge costituzionale, perché anche in audizione è emerso come pacifico il fatto che la procedura con la fiducia è una procedura speciale. Al di là di questo, quello che più mi sembra rilevante in questo momento, sul piano politico e non solo, è che ciò costituisce una clamorosa smentita delle dichiarazioni programmatiche su cui il Governo in carica ha ottenuto la fiducia nei due rami del Parlamento. Oggi ci troviamo con un comportamento che è in contrasto con le dichiarazioni programmatiche, senza che vi sia stata alcuna crisi di Governo e alcun cambiamento significativo. Il presidente presidente Gentiloni Silveri ha detto delle cose in Aula, che ora sta smentendo con il suo comportamento. Nel dibattito parlamentare sono emerse molte criticità. Si è parlato ad esempio dell'attribuzione dei seggi ad alcune Regioni a prescindere dal numero degli abitanti; delle deroghe introdotte per il Trentino-Alto Adige per garantire una minoranza linguistica, con un sistema che prevede che prevede criteri completamente diversi per l'assegnazione dei seggi. Lì c'è un sistema misto che è più maggioritario e meno proporzionale, anzi è sostanzialmente tutto maggioritario. Un altro aspetto lo ha appena illustrato il collega del mio Gruppo Fornaro.

contengono delle distorsioni che, secondo me e secondo noi, rendono il sistema incostituzionale. La prima osservazione che faccio (la meno grave, ma da questo dobbiamo partire) è che al cittadino non è offerta alcuna possibilità di esprimersi per il candidato uninominale. Il cittadino che non intende votare una lista non ha alcuna possibilità; il cittadino che è attratto dal nominativo che viene segnalato come candidato al collegio uninominale

o rinunciare al candidato che avrebbe votato o astenersi dal voto; e questo è in sé un elemento di una certa gravità. comprima in modo inaccettabile beni giuridici, cioè che contiene un'inaccettabile distorsione del voto del singolo cittadino, è il sistema di ripartizione del voto nel caso di più liste collegate. Il meccanismo è che io appongo il segno sul candidato all'uninominale e il mio voto viene trascinato sulla lista del proporzionale, quindi sul collegio plurinominale. Cosa vale il mio voto? Chi determina il peso del mio voto? Viene attribuito a qualcuno in particolare? Il peso del mio voto viene determinato dal voto che danno gli altri elettori nello stesso collegio. Quindi il peso del voto del singolo cittadino, che la Costituzione vuole diretto, eguale, libero e personale, libero e personale, dipenderà da come nel collegio vanno le cose, da chi nel collegio voterà in un modo o in un altro. Quindi la personalità del voto viene compromessa in maniera irreparabile.

Siamo nell'ambito dello stesso articolo 1, ma la medesima circostanza si verifica poi al Senato. Questa dicotomia sembra giustificata dal fatto che in un luogo si parla al cittadino e nell'altro luogo, invece, si parla della ripartizione dei voti. E anche questa differenza terminologica determina

del cittadino, secondo l'avvertenza che contiene la sua scheda elettorale, viene frazionato in più liste e, quindi, egli vota contestualmente liste con programmi e *leader* politici completamente diversi. Se questa interpretazione sembra fantasiosa, nonostante il tenore della legge, e se si vuole dire che i voti vengono messi in un calderone e poi insieme vengono distribuiti, allora si crea un sistema in cui il voto del cittadino andrà a una delle liste in maniera anonima: *tot, tot, tot*. Il mio voto andrà a una delle liste collegate e, in questo caso,

il voto, a chi potrà essere assegnato il suo voto, e anche questo incide sulla libertà e la personalità del voto stesso. Concludo con un altro elemento con un altro elemento che chi ha scritto queste norme ha tenuto in particolare considerazione. Si vuole dare una risposta possibile, dal punto di vista di chi ha scritto e votato queste regole, alle sentenze della Corte costituzionale, la n. 1 del 2014 e la n. 35 del 2017, che entrambe ribadiscono il principio della riconoscibilità. Anzi, forse in maniera più chiara la n. 35 del 2017 esplicita e commenta il contenuto della n. 1 del 2014. Le liste sono corte e, pertanto, non contengono il numero delle persone che dovranno essere

quando noi poi andremo alla ripartizione e alle liste e avremo davanti, eventualmente non una, ma due, tre o quattro liste, alle quali distribuire il voto o i voti, succederà

Quando però sarà dichiarata incostituzionale, ci saranno un altro *Premier*, un altro Ministro per i rapporti con il Parlamento e un altro Parlamento. Dunque, continuare su questa strada mi sembra un modo di procedere non certo da costituenti, che non segue neanche le regole della buona politica che mi hanno portato a sedermi in questi banchi. onorevoli cittadini che seguite i nostri lavori, il Presidente ha detto che i lavori in Commissione si sono svolti in maniera legittima, nel rispetto delle prerogative parlamentari, dal 17 al 23 ottobre.

mettere in sicurezza il sistema. Il vostro unico obiettivo è mettervi in sicurezza, salvare le vostre poltrone. Avete paura di una forza politica antisistema come quella che è arrivata qui nel 2013 e ha fatto tremare, forse, in più di un'occasione, le vostre poltrone, visto che oggi dovete correre ai ripari e, per mettere in sicurezza il sistema, varate una legge elettorale truffa, una legge liberticida, una legge creata esclusivamente per mettere in difficoltà il Movimento 5 Stelle. È questo, quello che avete fatto. Avete studiato questo disegno di legge a tavolino sulla base dei sondaggi, sulla base dei risultati possibili guardando i sondaggi, così come avevate fatto con l'Italicum. Peccato che poi i sondaggi sono cambiati. Pensavate di affossarci e invece con quella legge potevamo vincere e stravincere e allora cambiamola, perché non va bene, neanche corretta dalla Corte. Cambiamola in maniera tale da fare il possibile per mettere in sicurezza il sistema. Queste sono le parole chiave. Questo è il vostro unico obiettivo.

Quando il Governo mise la fiducia sulla legge elettorale truffa del 1953, il Presidente del Senato si dimise e con lui altri membri dell'Ufficio di Presidenza.

Ebbene, mi spiegate cos'è un collegio plurinominale se c'è un solo candidato? Avete sei collegi uninominali e un collegione uninominale complessivo di tutta la Regione. Ovviamente questo è ridicolo, e cosa comporterà

un mese prima. Sapremo nomi e cognomi in ordine alfabetico dei componenti del Parlamento, perché saranno scritti a tavolino. Tutti quelli che sono stati candidati saranno direttamente eletti; nomi e cognomi scritti a tavolino un mese prima. Mi ricorda tanto le elezioni farlocche della Provincia: avete agito sull'elettorato attivo, qui agite sull'elettorato passivo; in quel caso, con il voto dei singoli consiglieri sapete prima cosa voteranno; in questo caso, limitate il numero delle candidature - sì - perché gli elettori non possono votare nulla. Gli elettori non possono mettere la preferenza, ma possono scegliere ma possono scegliere non il candidato, ma solo un partito che deciderà nomi e cognomi di chi andrà a sedere sulle poltrone. Altro che giro magico. Avremo un bel quadratone magico di tutti gli amichetti di Renzi e Berlusconi che andranno a sedere in Parlamento, e anche di quelli di Salvini. Voi volete elettori ciechi, che devono stare semplicemente zitti e muti. Per questo domani manifesteremo con una benda sugli occhi qui davanti al Senato, per dire no a una legge elettorale che ci vuole ciechi. Fermatevi Fermatevi finché siete in tempo. Evitate l'ennesima brutta figura a questo Parlamento. Avete ottenuto le ultime due leggi elettorali incostituzionali e ne fate una terza. Con quale coraggio?

Due su due! E siete le stesse persone che c'erano allora, quando avete votato il Porcellum. Gira e rigira, siete sempre gli stessi. Evitateci quindi l'ennesima figuraccia e riportate, come chiediamo, il voto

è una legge elettorale sicuramente imperfetta, perché non esistono leggi elettorali perfette, ma non certo incostituzionale. E cerco di spiegarne le primo punto, le leggi elettorali possono essere approvate con il voto di fiducia? Con la fiducia era già stata approvata la cosiddetta legge truffa nel 1953, ma la questione è stata posta alla Consulta per il caso dell'Italicum, approvato dalla Camera con questo stesso strumento nel maggio del 2015. Ebbene: nella sentenza n. 35 di quest'anno la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i rilievi sollevatigli su questo punto per manifesta infondatezza. secondo punto riguarda le liste bloccate. Nel 2014 la Corte costituzionale ha sanzionato le liste lunghe e bloccate del Porcellum perché non idonee a favorire la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori e tali da rendere la disciplina - cito cito testualmente - «non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto». Il Rosatellum prevede che le liste abbiano al massimo quattro candidati: è un numero esiguo e, quindi, a mio parere, compatibile con i parametri costituzionali. terzo punto riguarda le pluricandidature. Nel Porcellum un singolo poteva essere candidato in ogni circoscrizione; con l'Italicum le candidature plurime sono state ridotte un massimo di dieci. Proprio analizzando i problemi di incostituzionalità dell'Italicum, la Consulta le ha dichiarate ammissibili. È stata invece cassata la possibilità per il parlamentare plurieletto di scegliere liberamente per il collegio preferito. A tal proposito, il Rosatellum prevede un meccanismo automatico: il collegio plurinominale di elezione sarà quello in cui la lista cui è collegato il candidato ha ricevuto meno voti. quarto punto riguarda l'indicazione del capo della forza politica, ovvero il famoso "uomo solo al comando". Come già il Porcellum e l'Italicum, il Rosatellum prevede che ogni lista indichi nel proprio programma elettorale il nome del *leader*. La Corte costituzionale non è mai stata interpellata sulla questione, ma è la legge stessa a dire che, nonostante questa indicazione, «restano ferme le prerogative del Presidente della Repubblica» in materia di nomina del Presidente del Consiglio. Quindi, si tratta di un'indicazione meramente politica, che non può avere alcun rilievo dal punto di vista costituzionale. Il quinto punto riguarda la ripartizione *pro quota* dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali. La modalità di voto "preferita" dalla nuova legge è l'espressione della propria volontà tramite un segno tracciato sul simbolo del partito prescelto. È ammesso però anche il voto in favore del solo candidato nel collegio uninominale. In quest'ultimo caso tutti i voti così espressi saranno ripartiti *pro quota* (in base alla forza elettorale) tra i partiti che sostengono il candidato nel collegio uninominale. Non è il primo caso di ripartizione *pro quota* dei voti nella storia delle leggi elettorali italiane: sempre *pro quota* avveniva infatti lo scorporo del Mattarellum e nessuno ha mai avuto a che ridire sulla legge che porta il nome dell'attuale Presidente della Repubblica. chi si oppone a questa legge ha denunciato la presunta incostituzionalità del Rosatellum per la mancanza del cosiddetto voto disgiunto. Mi sembra, però, una posizione insostenibile. In particolare, alcuni costituzionalisti hanno sostenuto che viola il principio costituzionale del voto libero il meccanismo in base al quale, se l'elettore barra solo il nome del candidato nel collegio uninominale, il suo voto si distribuisce, insieme agli altri analoghi al suo, sui partiti della coalizione che lo sostengono nella parte proporzionale. viene la richiesta, appunto, di possibilità di voto disgiunto, ossia la possibilità di votare un partito di un'altra coalizione, o almeno del doppio voto, e cioè la possibilità di votare il candidato del collegio senza che la scelta si riversi sui partiti collegati. Qui bisogna essere molto chiari: il termine "voto disgiunto" fin qui è stato sempre usato - appropriatamente - per la facoltà dell'elettore di votare un candidato sindaco (o Presidente di Regione) e una lista non legata a tale candidato. Ma una cosa è eleggere un sindaco o un Presidente di Regione; altra cosa è eleggere candidati per la composizione di una Camera, senza peraltro che il voto uninominale possa produrre alcuna maggioranza. Permettere un voto schizofrenico per le due Camere significherebbe favorire l'ingovernabilità. Dunque, il voto unico rientra pienamente nella logica di una legge che spinge a formare coalizioni, attraverso le quali i partiti decidono di partecipare alle elezioni. Il voto disgiunto violerebbe allora la prerogativa dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti

Il voto disgiunto, insomma, non è una scelta costituzionalmente obbligata. In realtà il Rosatellum distingue i due voti e si limita a proibire il voto incoerente e - come ho già ricordato - forme di collegamento, attraverso apparentamenti e scorpori, erano già presenti nel Mattarellum. riguarda i collegi uninominali. Essi sono costituzionali per espressa affermazione della Corte che, nella sentenza n. 1 del 2014, portava i collegi come esempio virtuoso per garantire il rapporto diretto tra eletto ed elettore. Per tutti questi motivi, il nostro Gruppo voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità. colleghi, questa legislatura riserva continue sorprese. Pensavamo ingenuamente che la lezione del 4 dicembre, meno di un anno fa, fosse servita a qualcosa e invece niente, siamo alle solite. È proprio complicato per questa maggioranza pensare di rispettare per una volta la Costituzione e di fare una legge elettorale a partire da quanto la Consulta ha stabilito nella sentenza del gennaio 2014, con la quale questo Parlamento è stato dichiarato illegittimo. Siamo dinanzi all'ennesima legge incostituzionale, una coazione a ripetere. È incostituzionale perché viene violato il diritto di vedere rispettata la propria manifestazione di volontà,

Vorrei partire proprio dal dovere civico. In questi anni nel nostro Paese la distanza tra cittadini e istituzioni, tra cittadini e politica è cresciuta così tanto che è venuto meno quel senso di appartenenza che faceva sentire ognuno parte dello Stato. I motivi sono tanti e tra questi vi sono sicuramente l'aver messo da parte l'interesse collettivo a vantaggio della tutela e del perseguimento solo degli interessi di parte; l'aver contribuito ad aumentare le diseguaglianze con politiche sbagliate, inseguendo austerità e liberismo sfrenato; l'aver contribuito a far sentire la politica non in grado di rappresentare e prendersi cura dei propri cittadini, ma solo come casta che difende i propri privilegi. E i cittadini hanno smesso di votare, perché non si sono più sentiti rappresentati; hanno smesso di esercitare quel dovere civico così sancito dalla Costituzione perché da troppi anche grazie a leggi elettorali palesemente incostituzionali, non è stata più rispettata la volontà degli elettori e non si è consentito di far svolgere il voto in modo libero, uguale e sereno. Il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica ha portato leggi elettorali per le quali il voto di molti cittadini è stato ignorato. Aver abbandonato il sistema proporzionale con l'introduzione di soglie di sbarramento e premi di maggioranza in nome della governabilità ha voluto dire stravolgere il voto e il valore del voto; ha voluto dire violare quel principio di uguaglianza del voto che così bene racconta l'articolo 48 della Costituzione. E anche il Rosatellum prosegue in quella direzione, a partire dal fatto che con un solo voto, come è stato ampiamente spiegato, con un'unica scheda si vota per il collegio uninominale e per la lista proporzionale. Dunque il voto di coloro che eleggeranno il candidato nel collegio uninominale varrà il doppio di quello di coloro che invece potranno sperare di far valere il proprio voto almeno sulla lista bloccata proporzionale. Negare il voto disgiunto, negare quindi di poter esprimere due voti diversi, negare il cosiddetto scorporo, cioè quei correttivi che furono introdotti nel Mattarellum proprio per rispettare l'uguaglianza del voto vuol dire che siamo palesemente dinanzi a un furto di legittimità costituzionale e a una negazione di uguaglianza. Io potrei decidere di votare il candidato nell'uninominale che conosco o che ho conosciuto in campagna elettorale - e questo salverebbe il valore aggiunto della scelta del collegio uninominale, utile anche a ricostruire quel rapporto tra cittadini ed elettori - e potrei poi decidere di votare al proporzionale per il partito nel cui programma mi riconosco. Qui l'elettore sceglie solo il partito e poi i candidati scelti dai partiti. Nessuna libertà di scelta, nessuna libertà di voto, nessuna uguaglianza. Siamo dinanzi all'ennesima compressione della democrazia, senza alcun rispetto della volontà del voto, con l'aggravante che tutto questo avviene a pochi mesi da quando gli italiani, con il voto del 4 dicembre, hanno bocciato una riforma antidemocratica e anticostituzionale. Ma evidentemente quel progetto, caratterizzato dall'accentramento dei dei poteri nelle mani di una sola figura, dell'ideologia dell'uomo solo al comando, che è stata l'impronta dello spirito riformista di questo Governo, non è stato abbandonato, nonostante le pessime *performance* di questa legislatura dalla buona scuola al *jobs act*. Questa legge elettorale, inoltre, abbandona alcuni cavalli di battaglia e sarebbe interessante capirne il motivo. Per anni avete raccontato che la governabilità poteva essere garantita solo da leggi elettorali che avrebbero dovuto far conoscere, alla chiusura immediata delle urne e dei seggi, chi fosse il vincitore, la sera stessa o la mattina dopo. E, per avere questo risultato, sarebbero state necessarie leggi utili per attribuire seggi con maggioranze chiare; leggi con premi di maggioranza e soglie di sbarramento atte a raddoppiare il valore del singolo voto; un sovradimensionamento del voto del voto e, ancora una volta, un furto di voto. Improvvisamente con il Rosatellum è scomparsa l'esigenza primaria della governabilità. Nessuno ne parla più, perché questa legge, così com'è pensata, fingendo di avvantaggiare le coalizioni e favorendo le finte coalizioni, avrà come unico obiettivo un sistema punitivo per chi non si piega alle politiche da inciucio e iperliberiste; consegnerà inspiegabilmente seggi alla destra, soprattutto al Nord, e consegnerà un quadro fuori dalle urne molto, molto frammentato, al punto che ci vorranno giorni prima di capire chi avrà vinto e come e quali maggioranze governeranno. È chiaro che il PD e il suo segretario pensino a un "Governissimo", magari con Forza Italia, ma non avete tenuto conto che il quadro politico e sociale del nostro Paese è profondamente cambiato. Questa legge rafforzerà molto il centrodestra, con il rischio di regalare loro il governo del Paese; oppure avremo un Governo vero di centrodestra, dove però voi del PD sarete il centro in ostaggio della destra. E, per come in questi anni avete sdoganato e realizzato le peggiori politiche della destra, a partire dai non funzionerà più nemmeno agitare ad arte la grande coalizione, il fronte della sinistra contro l'avanzata della destra o dei barbari. Non funziona più, perché i cittadini sono delusi e sfiduciati. Questa volta non basterà più schierarsi contro, ma sarà fondamentale raccontare quale idea di Governo si ha; come si costruisce una vera alternativa alle politiche neoliberiste che hanno impoverito soprattutto i ceti medi e aumentato le disuguaglianze; come si dà certezza di lavoro; come si garantiscono la sanità e l'istruzione pubblica gratuita. Quando la sinistra fa troppo la destra, alto è il rischio di essere considerati tutti uguali. E allora è preferibile scegliere l'originale. Con la totale scomposizione del nostro quadro politico, vorremmo avvisare tutti che cambia anche il voto nell'uninominale. Non siamo più nel 1994, quando si fronteggiavano due schieramenti; questa volta saranno almeno quattro. Dunque, la partita è tutta aperta. Non esisteranno più i seggi garantiti, perché si naviga in mare aperto, e questo vale per tutti, al punto che questa legge potrebbe rivelarsi un *boomerang*. Forse non avete valutato bene questo. In tempi di antipolitica, i candidati dei collegi uninominali con una campagna campagna elettorale molto legata al territorio e molto riconoscibile, potrebbero coinvolgere gli elettori e far prevalere la scelta del candidato uninominale su quella del partito. E, siccome non volete prevedere il voto disgiunto, il quadro potrebbe cambiare e riservare forti sorprese, soprattutto a voi del Il 14 settembre 2005, per evitare l'approvazione di quella legge elettorale che persino chi ne rivendica la paternità ha definito una porcata, Luciano Violante, a nome dell'allora centrosinistra, centrosinistra, citava esponenti di centrodestra che chiedevano al centrosinistra di non votare riforme a colpi di maggioranza. Riporto quanto è scritto sugli atti parlamentari: «Si violerebbe un principio di Costituzione reale in forza del quale le regole di vita democratica di un Paese vanno scritte con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, non potendo e non dovendo obbedire a interessi elettorali di parte». E Violante commentava: «Onorevoli colleghi, noi chiediamo un momento di coerenza tra ciò che avete scritto nella scorsa legislatura e ciò che oggi state per fare. Il tipo di progetto che voi

il viatico, una delle armi migliori offerte al populismo. Ora volete davvero ripetere lo stesso errore? Pensate che, sbagliando ancora, vi porterà consenso e vittorie elettorali? Non capite che questo Paese ha bisogno di rappresentare, prima di tutto, la sua complessità per affrontare i problemi che abbiamo di fronte? Non chiediamo autocritiche o di essere saggi. Se non volete essere saggi, almeno siate coerenti. Ma, se nemmeno volete essere coerenti, siate almeno furbi: vi state togliendo l'ultimo barlume di credibilità e, prima di cadere nel ridicolo, fermatevi perché questa sarebbe l'ennesima legge incostituzionale che eleggerà un ennesimo Parlamento illegittimo, in in violazione anche delle norme europee, come è stato ricordato. Aggiungo un'ultima cosa. È del tutto incomprensibile - mi rivolgo ai colleghi del Partito Democratico - perché abbiate scelto questa legge, che avrebbe potuto fare tranquillamente la destra, ma i suoi componenti - come vedete - non sono nemmeno presenti tra i banchi a difendere questo provvedimento di cui prenderanno i frutti, ma di cui voi vi assumerete tutte le responsabilità politiche. È del tutto incomprensibile e questa legge, oltre tutto, non vi garantirà nemmeno una sicura rielezione.

coglievo, su sua indicazione, un'altra delle tante aporie e, cioè, delle tante irrazionalità e aberrazioni che l'Atto Senato 2941 contempla. Nel caso di sostituzione forzata di un eletto in un collegio uninominale che cosa succederà? Facendo riferimento alla tradizione delle elezioni con sistemi uninominali maggioritari, si pensa che si va a nuove elezioni.

uno strascico, capaci di incidere su un collegio plurinominale relativo al collegio uninominale. Se però nel sistema uninominale vi è un rapporto di fiducia con quella persona Grazie può tranquillamente venir meno quel rapporto fiduciario e si potrebbe avere un risultato elettoralmente del tutto difforme, senza che si incida sul collegio plurinominale.

Se una legge può essere irrazionale, innanzitutto non è affatto giusta perché la giustizia è razionalità non è neanche coerente con i valori della nostra Carta costituzionale. Diceva un certo Meuccio Ruini, che qualcuno qui dovrebbe ricordare, che si vince quando si convince. Qual è la dimensione con cui noi esseri umani possiamo convincere altri esseri umani se non quella della parola che, comunicando, esprime razionalità, che è quello stesso valore che ci rende tutti uguali?

Proprio ieri mi è capitato (ma non sempre le cose avvengono a caso, anzi è vero il contrario) di riprendere un vecchio scambio tra Kant e Constant, quello in cui si ragiona sul rapporto tra verità e menzogna. Kant era considerato dai suoi contemporanei, anche da studiosi successivi, quel filosofo che, quasi da bacchettone e moralista, sosteneva che la politica dovesse essere soggetta a controllo da parte della morale attraverso l'intervento della razionalità del diritto. Parlamentari molto più bravi del sottoscritto (non voglio citare i presenti perché altrimenti farei torto a tanti), costituzionalisti come Valerio Onida (non Carneade, ma Valerio Onida, ex Presidente della Corte direttori di giornali, certamente non vicini alla parte politica che rappresento (vedi Paolo Mieli), hanno espressamente parlato di alterazione e manipolazione dell'intenzione di voto del cittadino. Noi ancora ci poniamo ci poniamo domande sulla presunta costituzionalità della legge, quando c'è evidentemente, palesemente, solarmente, cartesianamente la prova provata dell'irrazionalità della norma? In Commissione, quando si sono svolte le audizioni, tanti hanno sollevato argomentazioni forti, credibili e razionalmente convincenti sui difetti, le aporie e le fragilità di questa norma voglio qui ribadirle, per quanto non tutte. Tra queste vi è il voto congiunto, meccanismo che sembra violare il principio di uguaglianza. Chi è intervenuto prima di me, anche nell'illustrazione della pregiudiziale, ha ricordato a voi che siete gli artefici del Mattarellum che quando non avevate raggiunto tali livelli di perversione quantomeno avevate messo in salvaguardia il diritto dell'elettore di poter votare «A», rimanendo il suo voto solo e soltanto su «A» attraverso o il voto disgiunto o lo scorporo. Badate che queste sono eccezioni che noi abbiamo provato, proprio nel pomeriggio di ieri, a rimarcare attraverso i nostri interventi in fase emendativa della norma; ma come al solito, quando c'era la discussione generale, quando si doveva intervenire sul merito delle questioni, la maggioranza era totalmente assente.

Però, quando si tratta di votare, senza aver approfondito in discussione generale gli argomenti, puntualmente, come i funghi, spuntano tutte le manine, tutti gli arti superiori (sempre che siano superiori) dei colleghi della maggioranza e votano. E lo fanno naturalmente assecondando il parere negativo sia del relatore che del Governo, perché tutte le nostre proposte emendative sono state considerate assolutamente inaccettabili. voglio anche aggiungere una considerazione sull'eventualità che è prospettata da una delle ultimissime agenzie che sono state fatte girare

prossimo venerdì mattina, si arriva a un voto sulla fiducia così frettoloso e anticipato? Non ci vuole tanto a capirlo: c'è paura non tanto delle conseguenze di manifestazioni di piazza che si potrebbero svolgere oggi e domani pomeriggio qua fuori, quanto che vengano a ottenere quella giusta e doverosa la maggioranza - paradossalmente - è anche dall'altra parte. Infatti, quando si tratta di votare provvedimenti contro i cittadini elettori, si squaglia come neve al sole quel velo per cui, apparentemente, ci sono una maggioranza e una presunta opposizione e tutto torna chiaro e nitido. Voi non volete far sapere agli italiani che qui si sta consumando un ulteriore esempio di come il potere, quando non è democraticamente orientato, considera i cittadini. Noi abbiamo però il dovere, oltre che il diritto, di testimoniare. Tutto questo sta gradualmente, lentamente e faticosamente venendo fuori e tantissimi cittadini, a partire dalle prossime consultazioni in Sicilia

ragionando sulla pubblica amministrazione e sulla produzione legislativa inerente alla riorganizzazione della pubblica amministrazione, sottolineava come a Strasburgo e a Bruxelles le nostre leggi non venissero più neanche tradotte, perché, anche se tradotte, rimanevano incomprensibili. Se una legge, che dovrebbe essere uno strumento *erga omnes*

è una legge democratica? Il buon vecchio Kant, memore della lezione illuministica, diceva che il vero potere democratico fa le cose non nel segreto, ma in pubblico, perché non ha paura del confronto e del dialogo. Se voi ponete la voi ponete la fiducia addirittura questa sera, dimostrerete a tutti gli italiani che avete una fottutissima paura che aprano gli occhi.

poi sconfessato dai voti successivamente prodotti, del collega Walter Tocci in relazione alla questione di fiducia sul *jobs act*. *jobs act*. Mi rivolgo a quelle poche persone che potrebbero sentire un sussulto di coscienza a fronte di un'ennesima porcata che che probabilmente si consumerà a breve. Credo che sia nell'interesse di tutti salvaguardare le istituzioni. Voi ci accusate di essere populisti, ma voi siete demagoghi della peggior peggior specie. Vi ricordo che quando è l'istituzione a essere demagogica e a ricorrere all'ignoranza per sottomettere e subalternare, allora non c'è più democrazia ma soltanto un regime partitocratico.

con la sentenza n. 422 del 1995 (presidente Baldassarre), cassò quella norma, scrivendo chiaramente che essa era in contrasto con i parametri costituzionali, perché non è ammissibile una norma di legge che imponga, nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche, qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati.

il concetto delle quote, e, dopo una discussione approfondita (basta andare a vedere gli atti del Consiglio dei Ministri), venne scritto, nel nuovo articolo 51, che «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». da tutti nel senso dell'adozione di una serie di politiche attive per promuovere la partecipazione delle donne alla politica, per far sì che le donne siano presenti nelle liste, ma non assumendo e anzi esplicitamente eliminando ogni riferimento all'obbligo di proporre agli elettori liste bloccate in questa maniera. Mi è stato detto che, nel prosieguo, la giurisprudenza costituzionale si è modificata. Signor

la Corte nel ragionamento alla base della sentenza del 1995. Se io ho una donna bravissima in una circoscrizione e la metto capolista e poi ho un'altra donna altrettanto brava e la voglio mettere al secondo posto (visto che più di due è difficile che vengano eletti), per legge non lo posso fare: al secondo posto ci deve andare un uomo, qualsiasi uomo, anche il più inadatto e il più incapace deve prendere il posto della donna bravissima, o viceversa. mi ricordo il dramma del 1994 e la ricerca affannosa di candidature civetta; ricordo i drammi delle liste dove non potevano trovare collocazione persone che avevano un radicamento sul territorio. Ma la domanda che pongo è come si fa a riproporre la stessa identica norma, a pena di inammissibilità della lista, quando la sentenza del 1995 l'ha dichiarata palesemente incostituzionale e non c'è nessuna successiva sentenza della Corte costituzionale

So che questo intervento servirà a poco, ma lo lascio come testimonianza del fatto che quando la Corte costituzionale, che viene così spesso invocata, si esprime nella maniera più chiara assoluta le sue sentenze vengono stracciate. Non solo: vengono stracciate senza che successivamente vi sia alcuna modifica della Costituzione, né alcuna legge ordinaria, né alcuna sentenza successiva della Corte volto a

È possibile approvare qui un'altra norma che sicuramente, portata all'attenzione della Corte, verrà cassata insieme ad altre anomalie? È una domanda che faccio, sperando che il Governo o il relatore mi diano una risposta.

«questa Corte non può esimersi dal sottolineare che l'esito del *referendum* *ex* articolo 138 della Costituzione del 4 dicembre 2016 ha confermato un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive. In tale contesto, la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee». Lo dice la Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 e credo che sia il monito che avrebbe dovuto guidare la riflessione di tutti, arrivati a questo momento della situazione parlamentare e del dibattito parlamentare. Qualcuno in quest'Aula crede che con il Legalicum o il Consultellum si darebbe al Paese la possibilità di scegliere maggioranze stabili e omogenee? Si crede che con il Legalicum e il Consultellum davvero saremmo di fronte a un voto uguale e pari per tutti?

che, personalmente, non ritengo la legge migliore. Io avrei preferito una legge maggioritaria, davvero maggioritaria. Questa, però, è la legge e, di fronte a questa legge, per l'ennesima volta abbiamo assistito allo spettacolo del no *a priori* e del no che si succede su tutte le proposte di legge elettorale che vengono avanti, magari con la contraddizione nel senso che, per ciascuna legge, si usano quegli argomenti che nel caso precedente si sono utilizzati per il fine opposto. Detto questo, bisogna fare una distinzione, quando si parla di pregiudiziali di costituzionalità, tra quelli che sono profili riguardanti davvero il contrasto alla Costituzione e le questioni di "benaltrismo", cioè di preferenza per altri modelli. Questo "benaltrismo", che è lo sport più praticato, purtroppo è la dimostrazione, come in altre occasioni, di un'opposizione della pura critica distruttiva, fine a se stessa, per la quale va bene tutto e il contrario di tutto, purché non si arrivi a una soluzione. E che senso di responsabilità c'è quando ciò riguarda la legge elettorale, cioè quando riguarda le regole per la definizione delle Assemblee parlamentari? In questa prospettiva vi è una prima sottolineatura che mi sembra debba essere svolta. La nostra Costituzione disegna una Repubblica parlamentare, cioè incentrata sulla centralità del Parlamento senza investitura diretta del *Premier*. In questo contesto, come la storia insegna, sono compatibili modelli elettorali puramente proporzionali, modelli misti o modelli maggioritari. La scelta spetta al Parlamento nella sua amplissima e autonoma determinazione, senza che vi siano sistemi siano sistemi elettorali incostituzionali salvo, per l'appunto, quelli presidenziali o semipresidenziali. Ed è ciò che è avvenuto dopo il *referendum* degli anni Novanta su proporzionale e maggioritario, per responsabilità di una classe politica che non ha mai dato piena attuazione al risultato referendario e cioè al sistema maggioritario. Oggi il Senato è chiamato a votare un sistema maggioritario al 36 per cento e proporzionale al 64 che garantirà rappresentanza con lo sbarramento del 3 per cento e che non preclude la governabilità, come del resto il Mattarellum e il Porcellum, attentamente calibrati, diciamo la verità, per evitare l'effetto maggioritario pieno, tabù della classe politica degli ultimi vent'anni, vent'anni, impaurita da un sistema veramente maggioritario per amore del consociativismo. Nonostante questo, il sistema oggi all'esame viene accusato di essere incostituzionale perché non assicurerebbe né la rappresentanza, né la governabilità. In sostanza si vuole sostenere, sotto il primo profilo, che l'unico sistema ammissibile è il proporzionale puro. Nella Costituzione non è scritto. E l'esperienza degli Stati democratici ci dimostra che i che i correttivi a questo modello sono abbondantemente presenti, a partire della "mitica" Germania. Quale sarebbe, quindi, in una proposta come quella che emerge in questa legge, la norma costituzionale violata? Peraltro non vi è chi non veda la contraddizione di chi accusa queste leggi di non garantire la governabilità dopo aver urlato «al lupo, al lupo!» contro l'Italicum perché avrebbe garantito la governabilità e oggi denuncia l'incostituzionalità del disegno di legge al nostro esame perché non garantisce la governabilità. Una terza alternativa non è data ed è abbastanza singolare che oggi si invochi la governabilità come parametro di costituzionalità dopo avere sostenuto che la Costituzione garantisce la sola rappresentatività. È pacifico, in base alla giurisprudenza costituzionale, che il grado di governabilità proprio di una legge elettorale è rimesso alla discrezionalità del legislatore con il limite delle irragionevolezza e della illogicità manifesta, ed è evidente che in un sistema parlamentare le variabili possono essere molteplici. Tra queste rientra anche il Rosatellum 2.0 che si caratterizza per la commistione di due sistemi - proporzionale e maggioritario

introduce una strada che supera le molte critiche che in questi cinque anni sono venute ad un Parlamento che è depotenziato e cui è tolta la propria funzione. Ma le critiche che sono state portate a questo disegno di legge con le pregiudiziali sono naturalmente anche altre. Lascio stare quelle che non meritano considerazione, nel senso che appartengono ad una esasperata dialettica polemica che credo non faccia onore a questa Aula e che è il caso di non riproporre. Si è detto in primo luogo che si violerebbe l'articolo 48 della Costituzione perché il voto non sarebbe personale e diretto. Orbene, dal punto di vista costituzionale, il tema del rispetto dell'articolo 48 della Costituzione è legato ad una disciplina chiara dell'effetto del voto. Tale disciplina, in questa legge, è e, tanto perché sia ancora più chiara, è apposta sul retro della scheda, perché ciascun elettore possa decidere come votare e possa decidere se dare il voto tanto all'uninominale quanto al plurinominale o come diversamente comportarsi. Vi è un principio di voto unico, è una scelta è una scelta che nella Costituzione non trova un elemento di contrarietà. Si poteva scegliere un altro modello? Certamente, ma questo è il modello che è stato scelto e sottoposto. È una questione di scelta legislativa e di opportunità politica. Ma con la costituzionalità non ha nulla a che fare. Non è un caso che non si siano elencati elementi veri di incostituzionalità sotto questo profilo. Ci si è lamentati dell'eccesso delle soglie; ci si è lamentati della soglia dell'uno per cento, ma ho sentito anche in questa Aula osservazioni che ritenevano le soglie troppo alte perché disperdevano il voto sotto soglia.

del dieci per cento. È un principio che recupera democraticamente il voto degli elettori alla propria funzione. Ci si è lamentati anche della disciplina che prevede l'assegnazione dei seggi quando i quozienti non sono pieni o quando comunque si arriva a un punto per cui il seggio deve essere assegnato fuori dal proprio contesto. A questo proposito voglio leggere quanto dice la sentenza n. 35 del 2017: «Con riferimento al sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 se è costituzionalmente legittimo che il riparto di seggi avvenga a livello nazionale, (…) l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione deve essere quindi osservato fin tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere la legittimità di residuali ed inevitabili ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un'altra.

rimessa all'autonomia del legislatore. Dov'è il contrasto tra questa ipotesi e le norme che riguardano la legge costituzionale?

Presidente, colleghe e colleghi, chiedo un momento di attenzione. In mezzo ai lavori convulsi di questi giorni una pausa di riflessione può fare bene. Vorrei ricordare un evento di cui ricorre quest'anno il centenario. Il 24 ottobre, secondo il calendario giuliano, o il 7 novembre, secondo il calendario gregoriano, del 1917 esplodeva nel mondo la rivoluzione in Russia. Mi sono interrogato sull'opportunità di proporre qui, nel Senato della Repubblica, il ricordo di questa data; sono consapevole che questo può arrivare a turbare la sensibilità di alcuni e di alcune, che legittimamente possono nutrire nei confronti di quell'evento un'ostilità assoluta, ma siamo a cento anni da quella data e possiamo parlarne, come io intendo fare, con passione e nello stesso tempo con disincanto. Non so se è verità o leggenda, quella volta che chiesero a Chou en-Lai, anni Cinquanta del Novecento, che giudizio si sentisse di dare sulla Rivoluzione francese del 1789. E la risposta fu: «Troppo presto per parlarne». Di quei «dieci giorni che sconvolsero il mondo», secondo il *reportage* che ne fece il giornalista americano John Reed, trattano oggi molti giornali, molte riviste e molti libri. per mettere un pizzico di ironia in avvenimenti che hanno dalla loro parte non poco di vicende tragiche, si potrebbe dire che anche questa, come facciamo spesso in quest'Aula,è la commemorazione di un defunto: qui, a Palazzo Madama, come a Montecitorio, soprattutto nella I legislatura, seguita alla Costituente, presero posto alcuni protagonisti che avevano vissuto quella storia in prima persona. Questo mio ricordo vuole essere anche un omaggio a questi Padri. Il 1917 è conseguenza del 1914. Senza la Grande guerra non ci sarebbe stata la Grande rivoluzione. E la cosa da ricordare subito è che la prima rivendicazione, che forse più di altre produsse il successo della rivoluzione, fu la rivendicazione della pace: la pace ad ogni costo, si disse, anche a costo di perdere la guerra. Quando Lenin, contro tutti, firmò il Trattato di Brest-Litovsk, accettò tutte le più pesanti condizioni, pur di riportare a casa i soldati. Lenin era l'autore di quella che a mio parere è stata la più la più audace forma di appello rivoluzionario, quando disse

C'era quella idea, che era stata per prima di Marx, dell'internazionalismo proletario; un'idea niente affatto di parte, che affonda invece le sue lunghe radici nell'umanesimo moderno. Già nei moti rivoluzionari del 1905, i soldati si erano rifiutatati di sparare sulla folla e avevano sparato sui loro ufficiali; 1905 e 1917 sono le due tappe della rivoluzione in Russia. La lucida strategia, che sarà dei bolscevichi contro i menscevichi, era che i comunisti dovevano mettersi alla testa della rivoluzione democratica per portarla alle sue naturali conseguenze, che stavano nella rivoluzione socialista. Se democrazia è infatti il *kratos* in mano al *demos*, il potere in mano al popolo, quale strumento più democratico dei *soviet*, dei consigli degli operai e dei contadini? Ma, attenzione, i *soviet* dovevano farsi Stato, dovevano assumere l'interesse generale. E il fatto che invece di farsi Stato si sono fatti partito, chissà che non sia stato questo il vero punto di catastrofe dell'intero progetto. Ma comunque quella democrazia diretta non ha niente a che vedere con l'attuale democrazia immediata. Questa non solo non si fa istituzione, ma è antistituzionale e dunque antipolitica e allora è conservatrice, se non addirittura reazionaria. La rivoluzione partì su tre parole d'ordine: la pace, il pane, la terra e parole semplici, che toccarono il cuore dell'antico popolo russo; tre cose che erano state sottratte a quel popolo e la rivoluzione gliele restituì. Per questo l'assalto al cielo, che avevano già tentato invano gli eroici comunardi di Parigi, vinse a Pietrogrado con l'assalto al Palazzo d'Inverno. Colleghi, Presidente, conosco bene il seguito della storia. Una rivoluzione, che era nata dalla guerra, si trovò in guerra con il resto del mondo, accerchiata e combattuta. Non intendo, per questo, nascondere, tanto meno giustificare, le deviazioni, gli errori, la violenza, i veri e propri crimini commessi. Qui, c'è il grande problema del perché la rivoluzione, cioè il progetto di trasformazione in grande del corso della storia, sfocia storicamente nel terrore. E il problema non riguarda solo i proletari: i borghesi non hanno fatto di meno nelle loro rivoluzioni. La rivoluzione inglese di metà Seicento e la Rivoluzione francese di fine Settecento, ambedue hanno fatto cadere nel capestro la testa del re. E la Rivoluzione americana, per produrre la più stabile democrazia del mondo, è dovuta passare per una terribile guerra civile. Rivoluzione e guerra, dunque, rivoluzione e terrore sono inseparabili? Dobbiamo dunque, per questo, rassegnarci alla pratica di cosiddette pratica di cosiddette riforme graduali, che però mai riescono, minimamente, a mettere in discussione il rapporto - che poi è un rapporto di forza - tra il sotto e il sopra, tra il basso e l'alto della società? Questo è il problema che ci pone ancora oggi, dopo un secolo, quell'ottobre del '17. Ecco perché vorrei, se possibile, isolare il valore liberatorio di quell'atto rivoluzionario dai fallimenti epocali e anche dalle costrizioni antilibertarie, che lo hanno seguito nella sua realizzazione. Ricordo una data e condanno una sua successiva negazione. Quell'atto trova la sua fondazione nel mirabile inizio di secolo. Il primo decennio del Novecento vede l'irrompere, anch'esso sovversivo, della trasvalutazione di tutte le forme: in campo artistico, con le avanguardie, arti figurative, poesia, narrativa, musica; l'avanzare del principio di indeterminazione nelle scienze esatte e il crollo della meccanica newtoniana; nel pensiero filosofico, con la messa in questione della ragione illuministica. Come potevano le forme della politica, organizzazioni e istituzioni, non essere travolte da questo *Sturm und Drang*, da questo impeto e assalto? Come la grande Vienna è stata il cuore di quel sommovimento culturale, così Pietroburgo diventa il cuore di un sommovimento politico. Il secolo ne sarà interamente segnato. «L'anima e le forme» è lo splendido titolo di un libro del giovane Lukàcs, che esce nel 1911. Era l'anima dell'Europa ed era, come dirà anni dopo Husserl, la crisi delle scienze europee a ribaltare tutte le forme ottocentesche. Colleghi, lo spirito anticipa sempre la storia. La rivoluzione del '17, in Russia, sta in mezzo a questo totale fermento. Atto di liberazione, che metterà in moto masse enormi di popolo e provocherà scelte di vita di piccole e grandi personalità. Ad esso si richiamavano molti dei ribelli antifascisti, mentre subivano il carcere e l'esilio, molti dei combattenti nella guerra di Spagna contro i franchisti,

Se leggete le lettere dei condannati a morte della Resistenza, in Italia e in Europa, troverete spesso l'ultimo grido di saluto per quell'evento. Mi rendo conto di parlarne con fin troppa partecipazione e perfino troppa enfasi, ma vedete, colleghi, mi considero figlio di quella storia. Francamente, vi dico che non sarei nemmeno qui se non fossi partito da lì, qui a fare politica per gli stessi fini con altri mezzi, senza ripetere nulla di quel tempo lontano, passato attraverso tante trasformazioni, rimanendo però io stesso identico. Vi assicuro: è un esercizio addirittura spericolato, ma entusiasmante, se entusiasmo può esserci ancora concesso in questi tristi tempi. Vi chiedo ancora scusa.

desidero richiamare alcune evidenze legate alla celebrazione di questo centenario. La prima più grande evidenza è il fatto che la Rivoluzione russa

Ideologie che hanno sintetizzato un punto di vista sull'uomo molto semplice: il potere è tutto e l'uomo non è niente. Questo forse è il cuore vero di quella stagione ideologica perché l'ideologia è proprio questa capacità di rappresentazione della realtà in cui il mito dell'uomo nuovo trascende ampiamente i dati della realtà stessa e si arriva al cuore dell'uomo solo attraverso la scorciatoia della violenza. Quando Lenin e Stalin presero il potere in Russia, volevano creare una società su misura per gli operai e per i nuovi ceti proletari; ma la Russia non era quel Paese.

Così si sono regolati molti altri nella storia del Novecento. Nel «Mein Kampf» di Hitler, per molte pagine viene reiterata l'idea che l'uomo sia il perno di tutta la costruzione attorno alla quale far ruotare l'universo, ma da pagina 45 in poi Adolf Hitler scrive anche che gli ebrei non sono uomini e le conseguenze che trae sono figlie di quella logica. Quando Pol Pot, intellettuale che ha studiato alla Sorbona, torna nel suo Paese, decide di togliere la vita a coloro che portavano gli occhiali, perché se avevano gli occhiali potevano aver studiato qualcosa di diverso dal marxismo e per questo rappresentare la condanna dell'umanità.

una rivoluzione intesa come paradigma delle parole che citavo all'inizio: il potere è tutto e l'uomo non è niente. Oggi nuove ideologie fanno, con maggiore pervicacia, questo stesso raffronto: non è più la parola «popolo» ad essere presa in ostaggio, ma la parola «Dio». L'ideologia di matrice islamista, ad esempio, prendendo in ostaggio questa parola, rende sufficiente ancora poche ragioni per il proprio progetto di potere. Quello che dobbiamo imparare dall'esperienza della Rivoluzione d'ottobre, quindi, è che sempre, laddove l'ideologia ci prospetta il mito dell'uomo nuovo, questo conoscerà la sconfitta della realtà, cioè verrà inchiodato da quei dati di una umanità silente che continuamente è capace di interrogarci sul nostro destino, sul destino dell'uomo che è molto più grande della forza delle ideologie, perché la forza dei motori che muovono la storia si ritrova appunto nel cuore dell'uomo. Non potrò mai dimenticare aver imparato il senso della lotta alle ideologie da una trasmissione televisiva, che un uomo che siede su quei banchi ha riproposto a tutti noi: la trasmissione era «La notte della Repubblica», cioè la notte di una stagione in cui delle persone hanno dimenticato la propria umanità, proprio perché vinte e convinte da un'ideologia che li teneva in ostaggio. Spero che il ricordo che ci ha proposto il professor Tronti possa in questa circostanza ricordare a noi che la nostra umanità è più grande di tutte le forme che l'ideologia assume per farci dimenticare ciò che è vero, ciò che è bello e ciò che è giusto. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la votazione sulle questioni incidentali avrà luogo alle ore 17. Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 16,30.

Di Guido Rossi si è parlato molto dopo la sua scomparsa. E' stato detto da molti che era un grande giurista e un grande democratico,

nel suo studio di avvocato o a pranzo con amici, la sua intelligenza non si fermava mai, non smetteva mai di pensare, di progettare, di studiare e anche di sorridere, perché a Guido Rossi piacevano la buona conversazione, la letteratura, l'arte, la poesia, le cose ben fatte fatte e anche le persone perbene. Aveva uno sguardo veramente speciale, due occhi acutissimi che sprizzavano sempre interesse e curiosità; in quello sguardo c'era tutto, la sua intelligenza e la sua volontà, la sua allegria e la sua serietà. La ricchezza dei suoi interessi, la libertà di giudizio, la continua ricerca del nuovo non rendono facile catalogarlo negli schemi a cui siamo abituati: era certamente un giurista e un democratico, ma anche molto altro. Profondo conoscitore del nostro diritto, lo ha insegnato nelle più importanti università italiane, ma era anche un grande esperto degli ordinamenti giuridici delle democrazie occidentali e persino dell'intricata legislazione europea. È stato un grande avvocato, un professionista di talento a cui per decenni si sono rivolti i protagonisti dell'economia italiana chiedendogli aiuto per la soluzione delle questioni più intricate e difficili. Primo presidente della Consob, in quel ruolo è stato un vero servitore dello Stato. Ha governato la Consob con equilibrio, considerando tutta la delicatezza dell'attività di una istituzione pubblica indipendente che era chiamata a operare pionieristicamente in anni difficili e molto rischiosi. È stato senatore della Repubblica e la legge sulla concorrenza di cui è stato autore, in realtà per lui fu un importante tassello di un lungo lavoro che lo ha visto impegnato per tutta la vita nel tentativo di trasformare in una realtà trasparente, concorrenziale e pulita un mercato che lui giustamente vedeva opaco, segnato da epidemici conflitti d'interessi. È stato anche un autorevole capo azienda, chiamato a risanare importanti multinazionali colpite non solo da gravi crisi industriali e finanziarie, ma anche dalla perdita di parte della loro credibilità e onorabilità. Ripensando alla vita di Guido Rossi e alle straordinarie qualità che lo hanno portato a primeggiare ovunque, viene spontaneo domandarsi quali fossero i fili che univano in una sola persona un talento così vario, tanti interessi e così vivaci. È una domanda difficile anche per chi ha conosciuto Guido Rossi e gli è stato amico. Forse dobbiamo far passare un po' di tempo, almeno quello necessario a rileggere i suoi libri, i suoi scritti, a riflettere sulle sue posizioni pubbliche, a ripercorrerne la vita professionale ed istituzionale, a ripensare

ha sempre vissuto nella più assoluta linearità del pensiero e nella più completa correttezza dell'azione. Nella battaglia quotidiana tra il bene pubblico e l'egoismo della società possiamo dire che ha sempre combattuto per affermare la priorità dello Stato di diritto e delle regole dell'equità. A me piace pensare che una buona sintesi della personalità di Guido Rossi la si possa trovare nel suo rapporto con l'arte, la sua grande passione vissuta visitando mostre e musei, andando ovunque ci fosse qualcosa di bello che meritasse un viaggio o una visita. È stato un grande collezionista, molto rigoroso e attento alla coerenza culturale delle sue scelte. Guido Rossi, l'arte non l'ha soltanto guardata e ammirata, ma l'ha anche studiata in profondità, col rigore che metteva in tutte le cose cui teneva. Voleva capire fino in fondo il significato delle opere che guardava o che comprava, perché sapeva che solo così, solo capendole in profondità, avrebbe potuto amarle di un amore veramente consapevole. Gli piaceva ripetere una frase di un importante storico dell'arte veneta, suo grande amico, Alessandro Bettagno, che spesso diceva: «Nei quadri uno vede quello che sa». modo, un altro grande, Federico Zeri, completava il pensiero di Bettagno dicendo: «Il quadro costituisce una sorgente di conoscenza, piuttosto che di piacere». sono due espressioni magnifiche, perché sintetizzano con molta lucidità quanto la conoscenza e la cultura possano aiutarci a raggiungere il vero godimento dell'opera d'arte. Guido Rossi sapeva che qualsiasi grande opera, fosse quella di un surrealista o di un dada, ma anche un capolavoro dell'arte veneta del Settecento, o un prezioso libro del XVII o XVIII secolo, per essere veramente compresa e ammirata ha bisogno di essere guardata sapendone apprezzare il significato profondo, laddove sapere vuol dire non soltanto conoscere la storia e l'orizzonte culturale dell'opera, ma anche, come diceva Guido Rossi, arrivare in profondità, sino alla conoscenza delle tecniche e delle ricerche espressive ed estetiche che si sono susseguite nei secoli e hanno guidato la mano e la mente dell'autore del quadro. Ho ricordato tutto questo, perché penso che per Guido Rossi il bisogno di conoscenza non valesse solo come regola da seguire davanti a un quadro o in un museo. Per lui la sete di conoscenza è stata una regola di vita, un metodo con cui ha affrontato ogni capitolo della sua ricca esistenza. Anche per noi, che sediamo in Parlamento, se non vogliamo accontentarci di osservare la realtà con uno sguardo superficiale, ma pensiamo che serva saper capire ogni cosa in profondità, l'imperativo deve essere quello di cercare di vedere il mondo con gli occhi della conoscenza e dello studio. Guido Rossi non si è mai fermato alle apparenze, non si è mai accontentato del primo sguardo, ma ha speso tanta parte delle sue energie e del suo intelletto per capire veramente e riuscire a vedere sino in fondo il senso profondo delle cose e degli avvenimenti. Questo è il lascito di Guido Rossi di cui noi dobbiamo tener conto. Noi, senatrici e senatori, ci troviamo a decidere ogni giorno, con il nostro voto, se approvare o no un emendamento, se dire sì o no a una legge. In questa funzione siamo garantiti dalla Costituzione, che ci assicura una piena libertà di mandato. Questa grande libertà accresce di molto la nostra responsabilità e non dobbiamo sprecarla nel gioco degli interessi o nel commercio delle idee. Affinché possiamo usare bene la nostra piena libertà in Parlamento, Guido Rossi ci ha lasciato detto che ogni nostra decisione deve essere guidata oltre che dalla ragion politica, anche dalla conoscenza dello Stato e delle sue istituzioni, che è sempre molto faticoso raggiungere, ma che sola può portarci a separare quel che serve davvero al nostro Paese da quel che serve al nostro interesse particolare. *(Applausi

nella sua lunga carriera Guido Rossi, classe 1931, ha ricoperto diversi ruoli, tra cui presidente della Consob, senatore, presidente di Montedison e poi di Telecom. Guido Rossi ha fatto anche parte del consiglio di amministrazione dell'Inter. Quindi, si non indifferente, invidiabile, di persona capace e di sicuro affidamento. Nel 2006, dopo lo scandalo di Calciopoli, Guido Rossi è stato nominato commissario straordinario della FIGC. L'esperienza di commissario della Federcalcio ha fatto di lui, fotografato con la Coppa del mondo in mano nello stadio di Berlino, l'avvocato più famoso, ma - forse - anche il più odiato dai tifosi di alcune squadre. L'ultimo incarico del suo studio risale all'anno scorso, nella trattativa con i commissari straordinari dell'ILVA, Grazie

la concerneva. Correva già l'anno 1996 quando Emilio Riva fece ricorso a lui per l'arbitrato con l'IRI. Vista la sua rettitudine sotto certi aspetti, si deve per forza ricordare quando furono chiesti 800 miliardi di lire come ultima *tranche* dell'operazione e lui ne

Al di là delle cariche, Guido Rossi era tra i più conosciuti giuristi italiani e tra i massimi esperti di diritto societario. Nato a Milano ottantasei anni fa, dopo la laurea in giurisprudenza a Pavia, per il *master* aveva scelto Harvard, in tempi in cui non era certo frequente che un giovane potesse andare a studiare in America. «Genio con la faccia da macellaio», lo definì Vittorio Feltri, rilevando che il professore sta a sinistra perché «lì le strade sono in discesa e Rossi non prende mai le strade Salvo poi aggiungere: «Non dirò mai una parola storta su di lui, perché la storia della sua famiglia mi incanta e mi commuove: figlio di un'impiegata del Comune di Milano, che l'ha saputo educare come chiunque di noi sogna di educare la prole. Il padre non l'ha mai riconosciuto, ma gli ha fornito i mezzi per laurearsi. Mai soldi furono spesi meglio». La sua fama di fenomeno comincia al Ghisleri, collegio di Pavia, officina di cervelli poveri, ma ambiziosi; si laurea poi in filosofia con una tesi su Max Weber. Weber. Rossi invece primeggia a giurisprudenza, tant'è che, ricorda un compagno di corso, «era lui a insegnare ai professori, non viceversa». Si era infatti laureato anni. Io non l'ho mai conosciuto, se non per questioni legate all'ILVA, e per questo mi sono permesso di fare quest'accenno. Guido Rossi è stato tra l'altro autore di diverse pubblicazioni, tra cui «Persona giuridica, proprietà e rischio d'impresa», «Capitalismo opaco», «Il mercato d'azzardo» Noi della Lega lo ricordiamo così, con questo piccolo intervento, facendo le condoglianze, anche se dopo qualche tempo, a tutta la famiglia.

allievo a maestro, di collaborare con lui per alcune delicate questioni. Non ho alcun bisogno di tratteggiare la sua maestria nel diritto:

Ma devo ricordare alcuni tratti umani di straordinaria levatura, che ho avuto occasione, insieme a mio fratello Nicola, di rilevare in lui. Il primo, lo ricordo con attenzione: di fronte a un atto stilato da un giovane avvocato del Sud, il professor Guido Rossi non si esercitava nel correggerlo profondamente, ma gli bastavano alcuni brevi tratteggi per approfondire le questioni essenziali, coglierne i punti giuridici di fondo e talvolta innovare profondamente sul diritto esistente o vigente a quell'epoca. Egli è stato infatti, per alcune questioni del diritto commerciale in Italia, un vero e proprio innovatore. Le sue opinioni, a lungo dibattute in dottrina e in giurisprudenza, si sono poi affermate e consolidate definitivamente nell'ordinamento. Conservo ancora alcune delle sue brevi correzioni, molto puntuali, approfondite e determinate. Il secondo aspetto che devo ricordare di lui è il rapporto profondo che aveva con la cultura. Mi raccontava sempre

Milano, nel primo dopoguerra, vi erano tre borse di studio annue che le potenze vincitrici avevano stanziato in favore delle potenze sconfitte: Italia, Germania e Giappone. L'anno in cui il professor Rossi si laureò

giovane Guido Rossi, venne ammesso in maniera eccezionale e straordinaria a questo corso. Non a caso, infatti, quella sua formazione, consentì alla sua cultura giuridica anche una profonda

prima di tutto un grande esperto del diritto, un professore, un avvocato e poi anche un senatore della Repubblica. A nome mio personale e di tutto il Senato mi unisco al cordoglio dei senatori intervenuti e invito l'Assemblea a osservare un momento di riflessione e di silenzio.

prima di passare al voto delle questioni incidentali, avverto che la senatrice De Petris, a nome del prescritto numero di senatori, ha chiesto di votare a scrutinio segreto alcuni paragrafi delle premesse e del dispositivo della questione pregiudiziale QP2, in materia di minoranze linguistiche. La richiesta è inammissibile per le seguenti ragioni. Innanzitutto, l'articolo 93, comma 5, del Regolamento stabilisce che sulle questioni pregiudiziali e sospensive il voto «ha luogo per alzata di mano», quindi sono escluse le votazioni con procedimento elettronico (nominali o segrete). In particolare, la richiesta riguarda solo alcuni periodi della questione pregiudiziale QP2 e pertanto l'eventuale votazione a scrutinio segreto dovrebbe essere preceduta da una pronuncia dell'Assemblea sul voto per parti separate, anch'esso non praticabile su una questione incidentale. Infatti, il richiamato comma 5 dell'articolo 93 del Regolamento prevede che su tutte le questioni pregiudiziali - in questo caso quattro anche se sollevate «con proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione». La richiesta pertanto non può essere accolta.

Grazie Grazie

tutela il voto relativo alle minoranze linguistiche. Si parla di qualunque tipo di deliberazione, non si specifica voto di emendamenti, articoli o altro. Si parla di una deliberazione in senso lato. Pertanto, siamo di fronte ad una decisione su cosa

avvengano con scrutinio segreto - tutte, nessuna esclusa - questo prevale su ogni altra considerazione, in quanto è una materia disciplinata in maniera specifica e diretta. Dunque, non è possibile nemmeno interpretare qualcosa che nel Regolamento è già chiaro. Non si sta parlando di una Presidente, insisto, lei ha commesso una imprecisione nel rimandare a una successiva verifica ciò che è già chiaro e prescrittivo nel Regolamento vigente. Stiamo parlando di una legge elettorale; siamo in una fase in cui si vota per alzata di mano sulle questioni pregiudiziali e sospensiva. Il fatto che siamo su una legge elettorale raccomanda un pedissequo rispetto del Regolamento e non viceversa, non una flessibilità interpretativa. Ne abbiamo già viste tante qui: sulla riforma costituzionale, sulla precedente porcata incostituzionale dell'Italicum,

ringrazio i colleghi del Movimento 5 Stelle per la particolare attenzione ultimamente rivolta alle problematiche delle minoranze linguistiche.

Vorrei ricordare, come premessa, al senatore Zeller che il disegno di legge di cui stiamo parlando prevede un collegio proporzionale mascherato perché il collegio plurinominale per l'elezione di un solo candidato è sostanzialmente un maggioritario; a maggior ragione in una Provincia autonoma con il 70

è molto chiaro che qui dentro ormai sono saltate le regole così come i principi fondamentali del rispetto; sono saltate le procedure, è saltato il rispetto del dibattito. Perché il senatore Zeller non è venuto in Commissione Abbiamo discusso nel loro vuoto pneumatico. Perché non ha partecipato e non si è espresso perché si potesse discutere questa che è una stortura puntuale e macroscopica nello stesso tempo? Per quanto riguarda le questioni incidentali, l'articolo 93 del Regolamento è intitolato «Questioni pregiudiziali e sospensiva». Sono due materie distinte.

Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del disegno di legge n. 2941, recante: «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali», nel testo licenziato dalla Commissione, identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Grazie

Presidente, richiamo la sua attenzione sull'ordine dei lavori in quest'Assemblea. Siamo stati gravemente preceduti da violazioni dei basilari principi di rispetto istituzionale, non solo tra Gruppi parlamentari, ma anche verso i cittadini. Alla Camera dei deputati la legge elettorale, approdata in Aula, è stata rimandata in Commissione dopo che un sacrosanto emendamento che stabiliva la parità tra tutti i cittadini sul territorio italiano, e non una zona franca

minimo dell'Assemblea. Arrivato qui al Senato, il provvedimento ha avuto le ore contate. In Commissione è stato disposto un calendario compresso. Abbiamo subito l'affronto

torni sui suoi passi, consentendo la discussione generale e ponendo eventualmente la questione di fiducia, se, in base ai contenuti emersi, non deciderà - spontaneamente o "spintaneamente" - di ravvedersi su questo proposito. La discussione generale qui è sacra:

favore! La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4

all'organizzazione dei lavori sulle cinque questioni di fiducia poste dal Governo sull'approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del disegno di legge di riforma elettorale. La discussione unica sul complesso delle cinque fiducie, per le quali i tempi sono stati ripartiti in base a specifiche richieste dei Gruppi, inizierà oggi pomeriggio fino alle ore 21 e proseguirà domani mattina con inizio della seduta alle ore 9 e fino alle ore 14. La prima chiama, riferita all'articolo 1, avrà pertanto luogo a partire dalle ore 14, la seconda chiama (articolo 2) alle ore 15, la terza chiama (articolo 3) alle ore 16, la quarta chiama (articolo 4) alle ore 17. Alle ore 18 sarà votato ordinariamente l'articolo 5, sul quale non è stata posta la questione di fiducia. Seguirà immediatamente la quinta ed ultima chiama, riferita all'articolo 6. Le dichiarazioni di voto avranno luogo giovedì mattina, a partire dalle ore 9,30. Seguirà quindi il voto finale sul disegno di legge, orientativamente alle ore 11. Subito dopo si riunirà la Conferenza dei Capigruppo, per stabilire il calendario dei lavori delle prossime settimane.

il rispetto minimo delle regole non è solo un atto dovuto. Davanti ad un atto così, che non posso che qualificare

non solo per esprimere un giudizio ma per fare, signor Presidente, il proprio dovere. Tra l'altro, nel caso specifico i Capigruppo - come lei sa perfettamente meglio di me - hanno la possibilità di intervenire sull'ordine dei lavori.

Non c'è stata la possibilità, come si è visto, se non di illustrare le pregiudiziali e di fare un intervento per Gruppo. Questo è quello che è toccato al Senato toccato al Senato di discussione, quanto a possibilità per ogni senatore di poter dire la propria su questo disegno di legge, sulla legge elettorale, Presidente. Io richiamo qui, ancora una volta, l'articolo 72 della Costituzione. Vi sembra questa una procedura ordinaria? Questo è ordinario? Capisco che voi ormai siete abituati - lo dico ai rappresentanti del Governo - e che pensate che l'ordinaria amministrazione sia quella di votare tutto con la fiducia. Ma ci sono dei limiti che non si possono valicare, ci sono dei limiti alla decenza. Eppure l'avete visto con la riforma costituzionale: il Paese vi ha detto che non era d'accordo né nel merito, né nel metodo che avete usato. Ma questo non vi è servito di lezione. E dopo tutto questo siamo arrivati al punto, signor Presidente, che anche la discussione generale viene bypassata, perché facevate fatica anche a dover sentire qualche senatore che voleva esprimere il proprio giudizio e voleva fare il proprio mestiere. proprio mestiere. Per che cosa siamo stati eletti qua dentro, se non per dire quello che pensiamo, per esprimere un giudizio, per fare il nostro dovere? E il nostro dovere, in un Parlamento, è anche anche quello di intervenire! Noi non siamo abituati a obbedir tacendo, ma questo è diventato il nuovo *slogan* di quest'Assemblea. Questa, signor Presidente, sarà ancora una volta un'onta,

Di questo passo, sulla legge elettorale, in quest'Aula dobbiamo andare a elemosinare i tempi per potere intervenire sulla fiducia, perché in teoria si discute sulla fiducia, e non nel merito della legge! Questo è ciò che tocca a questo Senato! Signor Presidente, lei si deve ricordare che i cittadini italiani hanno detto che il Senato doveva continuare a esistere.

quest'Aula. Ancora una volta, purtroppo, si sta scrivendo un'orribile pagina nella storia di questa disgraziata legislatura, perché alla fine è stata una disgraziata legislatura. Solo colpi di mano! Questa è la sintesi di questa legislatura!

il fatto di poter discutere sulla fiducia al Governo non sana il *vulnus* della cancellazione della discussione generale nel merito del provvedimento. Questa è una ferita gravissima, perché è necessario distinguere l'oggetto. Una cosa sono i contenuti della legge elettorale e le distorsioni che infliggerà nell'espressione della volontà popolare; altra cosa è che un Governo chieda la fiducia, che è altra violazione, altrettanto grave di quello che dovrebbe essere, invece, il normale

si voterà la fiducia sull'articolo 6. Con ciò lei ha espresso, in modo informale, un punto evidente a tutti: cioè che la fiducia non è il voto normale per una legge elettorale. Dovevano essere separate le discussioni: una nel merito e l'altra sul metodo. Sul metodo, voglio far notare che abbiamo un Governo renitente rispetto a un obbligo previsto dalla legge di contabilità: cioè che entro il 20 ottobre sia presentata la legge di bilancio. Abbiamo un decreto fiscale, già vigente e strettamente connesso a questa legge, che richiede che s'intervenga e che questo Parlamento sia attivato per una una disposizione che è fondamentale, non solo per le casse dello Stato ma per tanti cittadini e imprese che si aspetterebbero soluzioni. Ebbene, noi abbiamo anteposto una legge elettorale di chiaro patteggiamento tra parti a dispetto dell'interesse nazionale sia rispetto alla volontà dei cittadini che hanno diritto di esprimersi alle urne sia rispetto all'urgenza che hanno i provvedimenti di natura economica e finanziaria. finanziaria. A questo Governo noi dovremmo dare la fiducia. La dobbiamo dare in una discussione sulla fiducia a pacchetto. Questo compromette la possibilità dei cittadini di comprendere ciò che sta avvenendo nelle Aule. Aule. Ripeto che il *vulnus* da questo punto di vista non si sana con la concessione di un tempo di discussione relativamente ampio (relativamente rispetto a precedenti situazioni). Anche se, trattandosi di cinque fiducie diverse, poste in maniera diversa sui diversi articoli, dovremmo pensare che ognuna riapra una questione e che ognuna vada discussa separatamente, come avevo chiesto. Diversamente, il Governo avrebbe potuto porre un'unica questione di fiducia su tutto il provvedimento. Noi sappiamo, però, qual è il vero motivo per cui questo non è stato fatto: non è stato fatto: perché avrebbe comportato una variazione nell'articolato e avrebbe portato di nuovo alla Camera il provvedimento, arrivando a doverlo votare in quella sede dopo le elezioni siciliane, che sono fondamentali. A questo punto, i siciliani sanno di avere nelle loro mani uno strumento importantissimo per modificare non solo la politica della loro Regione ma anche la politica italiana e di dare un calcio, definitivamente, a questa disgraziata legislatura, a questa maggioranza contro natura, a questo Governo fallimentare. Ecco, avremmo voluto, e ne avremmo avuto il diritto, che le discussioni nel merito della legge e sui sui metodi del Governo, che qualcun altro ha avvicinato ad esperienze di anni bui, di un ventennio che pensavamo finito, fossero separate. A questo punto allora, dopo avere rimarcato con la pacatezza

Rimarcati questi punti di cui deve rimanere traccia, relativi a quel che è avvenuto in quest'Aula, io sono a chiederle, Presidente, come atto dovuto, la pubblicità dei lavori attraverso la ripresa diretta quantomeno dei lavori in Aula di giovedì mattina, cioè le dichiarazioni di voto e il voto finale. finestra"). La Presidenza, nulla osservandosi in contrario, concede la diretta televisiva per le dichiarazioni di voto di giovedì mattina, che si svolgeranno a partire dalle ore 9,30. aperta la discussione congiunta sulle questioni di fiducia poste dal Governo sull'approvazione, senza modifiche, degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del disegno di legge n. 2941, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

quindi dovrei cambiare completamente il testo dell'intervento visto che il Governo, ancora una volta, ha usurpato la funzione del Parlamento, dimenticandosi che è un Esecutivo e quindi imponendo la sua volontà a tutti i senatori qui presenti che invece rappresentano il popolo, a differenza del Governo,

In questi quattro anni e mezzo ho avuto modo di veder superare tante volte i limiti, così tante volte che ormai ho perso il conto. Ed è ancora peggio se penso che prima di questa legislatura e ancora prima voi, e sempre voi, eravate qui a garantire questa assurda difesa del sistema. Ma per me che sono campano la parola «sistema» ha un significato ben preciso e tutti i presenti qua dentro sanno qual è quel significato.

Berlusconi e Salvini. Un accordo ovviamente di facciata che durerà il tempo di far emergere il vero protagonista di questa ennesima porcata fatta alle spalle dei cittadini. Il vero protagonista dell'accordo con il partito di Berlusconi è Matteo Renzi, sempre lui. Lui, il segretario del PD, che si è allontanato da Roma, lasciando ai suoi l'obiettivo di portare a casa il risultato in cambio di un posto in Parlamento. Anche questo, rasenta il ridicolo. Colui che aveva sostenuto che, perso il *referendum* costituzionale, sarebbe sparito dalla scena politica,

A voi, senatori del Partito Democratico, chiedo: avete la necessità di prostituirvi davanti al vostro capo Renzi per avere assicurato un posto? Questo è ciò che fate?

Una volta vi chiesi di ribellarvi. Voi non solo non l'avete fatto ma continuate ad essere schiavi delle catene che vi siete messi da soli. Sarete ancora schiavi di gente come Clemente Mastella! Nel sistema che avete proposto - per andare sul tecnico - ci sono *vulnus* democratici rilevanti. Ne dico solo due, Presidente: il primo è relativo alle soglie di sbarramento. Dite che c'è una soglia di sbarramento al tre per cento ma è una falsità.

Inoltre, con il meccanismo tramite cui il voto dato al candidato uninominale vale anche per le liste, la soglia non è dell'uno per cento ma ancora più bassa. Ciò significa che anche microscopici gruppi di interesse specifico - li potremmo chiamare i lobbisti del voto, i lobbisti di questa strana democrazia contribuiranno alle sorti delle ammucchiate coalizzate, perché queste sono: ammucchiate. Politicamente come spiegherete questa scelta, se non con la volontà di raschiare il fondo del barile? Il secondo e ultimo aspetto riguarda i programmi elettorali, questa cosa per voi sconosciuta. Il Movimento 5 Stelle sta lavorando da un anno alla scrittura di un programma per l'Italia, scritto con i cittadini e che sarà il nostro unico, vero biglietto da visita; l'unica cosa che ha davvero importanza, quello che dobbiamo fare per risollevare le sorti di questo Paese. Presenteremo questo programma e se gli italiani sceglieranno il Movimento 5 Stelle avranno la sicurezza che quel programma sarò messo in atto. Che cosa presentate voi invece agli italiani? Un'ammucchiata di liste in contraddizione tra di loro che serviranno solo come specchietto per le allodole, ma gli italiani non sono allodole e hanno la schiena dritta e ve lo dimostreranno. Gli italiani! Io voglio che i cittadini qui fuori ascoltino bene. Quale programma verrà attuato da Renzi con Salvini, con Berlusconi, con Alfano, con Verdini (e chi più ne ha più ne metta)? Come potranno convivere gli animalisti con i cacciatori? Gli ambientalisti con i trivellatori? A questo punto concludo, Presidente, rivolgendo un appello ai cittadini: abbiamo bisogno di voi; vi chiediamo di manifestare con noi, pacificamente, per far sentire la vostra voce. Vi chiediamo di portare

Abbiamo visto occupare lo scranno della seconda carica dello Stato.

Presidente, ho assistito al dibattito sulle questioni e mi accorgo con dispiacere che tutte le vostre argomentazioni, seppur sensate, non vengono prese in considerazione da nessuna parte. allora se «pregiudiziali» non sia un termine che viene dal giudizio preventivo, ma da un pregiudizio che avete come parti politiche e non come singoli che espongono le proprio idee e i propri ragionamenti. La mancanza assoluta di ascolto da parte del Governo sta a significare che la pregiudiziale di costituzionalità presentata in quest'Assemblea è solo un passaggio rituale che rischia di essere inutile. Magari un domani la Corte costituzionale ripeterà le medesime argomentazioni per cassare questa legge elettorale e tutti si stupiranno. Cominciamo dal 2013. Io, ma anche voi, voi, sono stata eletta con una legge dichiarata parzialmente incostituzionale, ma da va sé che il compito di questa legislatura sia solo - o sarebbe prudenzialmente dovuto essere - di ordinaria amministrazione. Così si esprime la Corte: ordinaria amministrazione. Questi cinque anni avremmo dovuto fare questo, ordinaria amministrazione. In fondo, cosa abbiamo fatto davvero finora di ordinario? Nulla. Quasi nulla. Poche leggi, magari vuote, come l'ultima sulla lingua dei segni, un provvedimento pieno di belle parole e principi, ma senza un euro per favorire la vera e piena integrazione delle persone sorde o sordocieche. Dimenticavo il capolavoro del Governo Renzi, la riforma del codice degli appalti; una riforma scritta con i piedi, che ha complicato la vita delle nostre imprese oneste e ha favorito il caos a vantaggio di quelle poco trasparenti. Questa grande riforma del Governo Renzi è giunta sul filo di lana della scadenza dei termini imposti dall'Europa, ma ha già subito l'onta di ben due decreti di *errata corrige*, di cui il primo con ben 180 correzioni, non solo formali. E le imprese che già arrancano sotto il peso di una burocrazia elefantiaca vi dicono grazie.

emanato un decreto-legge fiscale, che nasconde balzelli e nuove tasse, che non avete il coraggio di far emergere nella legge di bilancio, che invece riempite di marchette,

Avete ancor più toccato il fondo con le varie misure sulle banche, che hanno visto migliaia di piccoli risparmiatori privati risparmi di una vita, mentre i colpevoli dei vari *crack* bancari sono ancora a piede libero. Volevate risanare il sistema, ma non avete neppure avuto il coraggio di fare una vera Commissione d'inchiesta. È solo lo spauracchio di una Commissione d'inchiesta. Poi abbiamo assistito al becero tentativo di riforma costituzionale e ricordo che avremmo dovuto fare cinque anni di ordinaria amministrazione. Quindi, questo tentativo di riforma costituzionale, che ha impegnato il Parlamento per innumerevoli mesi, con conseguenti costi per i cittadini, cittadini, è fortunatamente fallito il 4 dicembre, grazie ad uno scatto di orgoglio degli italiani, che hanno respinto al mittente una legge costituzionale scritta male.

e che legge elettorale! Che cos'è una legge elettorale? La legge elettorale è quella

La legge elettorale deve essere frutto di un processo sano e democratico, anche di un ragionamento complesso, ma non deve produrre una norma criptica, a vantaggio dell'una o dell'altra parte, e a discapito del non più decidente popolo italiano. Essa è la legge fondamentale, che regola la democrazia del Paese. Possono esserci anche dei contrasti molto accesi attorno ad un tema, ma qui siamo in Parlamento e occorrono rispetto e dialogo, ma purtroppo oggi, qui, non vedo nessuno dei due: non vedo il rispetto e non vedo il dialogo. Non esistono il giusto e lo sbagliato, ma esistono obiettivi e criteri di priorità diversi, secondo i quali perseguire un bene comune. Se l'obiettivo di questa legge fosse stato deciso nel rispetto di tutti e con obiettivi chiari, non avremmo dubbi sul votarla e tutti potremmo decidere, in nome di quella che i nostri avi chiamarono democrazia, decidendo di votare la legge elettorale migliore

che, intenti a riposizionarvi ognuno al proprio posto, state lasciando via libera al male assoluto. La mancanza di rispetto e la mancanza di dialogo sono il male assoluto. Il non poter decidere insieme, il non poter votare insieme danno via libera al male assoluto. Sembra siate protesi verso il solo e avido desiderio di gestire il potere, senza avere nessuna capacità di valutare a chi realmente stiamo dando le redini del potere. State guardando il vostro cavallo di Troia e io assisto impotente a questo fatto. Mi dispiace che saranno cassati i miei emendamenti, che proponevano una cosa moderna: il voto elettronico. Tutti silenziosi, mesti, obbedienti, a tutti quanti auguro veramente un buon "ri-scranno", ma

Signor Presidente, colleghi, la discussione di oggi rappresenta un momento significativo di questa legislatura non soltanto per l'oggetto stesso del provvedimento, ma anche perché le discussioni correlate e alcune modifiche apportate sono la metafora più eloquente del momento politico e delle superficialità argomentative che lo stanno caratterizzando, ma queste premesse conducono anche ad altre riflessioni. La legge elettorale nasce da una premessa chiara a tutti: l'urgenza di armonizzare due schemi per Camera e Senato e di superare il Consultellum al fine di fornire un quadro applicativo chiaro non solo per lo scenario politico, ma anche per gli elettori. L'importanza di questo testo si colloca dunque ben oltre l'urgenza di riformare la legge elettorale preesistente, che ha condotto ad esperienze politico-governative che non necessitano di essere ulteriormente commentate. La priorità era creare una legge elettorale lì dove - nei fatti - mancava. Come si potrebbe essere contrari, oggettivamente, a questo principio? Pertanto sono sempre stato dell'idea che fosse urgente approvare in tempi rapidi una legge elettorale assolutamente necessaria, anche perché i tempi impongono sintesi e ordine,

caratterizzata anche da un certo logoramento delle posizioni. Del resto, se ad un'analisi di insieme non si può eccepire nulla circa la legittimità di un intervento sistemico di tipo elettorale a pochi mesi dalla scadenza della legislatura, si fa certamente più fatica a comprendere perché un intervento legislativo di urgenza - quasi tamponativo - debba diventare veicolo di riforme molto più complesse rispetto a quanto concordato. Questa leggerezza rischia di rendere, per certi versi, insensata la legge stessa, compromettendone un'originaria validità. Mi soffermo, per chiarezza, sull'incursione sull'incursione a sorpresa nelle norme che regolano l'esercizio di voto nella circoscrizione estero, di cui anche a livello mediatico si è discusso abbastanza. limitati ad inquadrare gli emendamenti correlati ad una sorta di cambiale, svilendo poi di fatto tutto il resto, si tratta di una disciplina complessa, per chi non lo sapesse, oggetto di una istruttoria nel 2001. Non voglio dilungarmi sul significato del voto all'estero, ma non posso esimermi dal definirlo un punto di approdo di un percorso di consapevolezza e di autocoscienza storica, sociale e politica durato decenni, che ha ristabilito equilibri di reciproca conoscenza ed attenzione tra cittadini dentro e fuori i confini nazionali, conducendo il nostro Paese, dopo decenni di massiva emigrazione, a fare i conti con la propria storia. legge Tremaglia non è un semplice ventaglio di norme: è prima di tutto un percorso storico-politico che ha condotto ad una riforma costituzionale con una sua *ratio*, e che a distanza di appena sedici anni sembra che il Parlamento abbia già rimosso. Quanto contenuto nell'articolo 6 del disegno di legge in esame non è affatto residuale, ma determinante. Il superamento del vincolo della residenza nella circoscrizione estero per i candidati è qualcosa di più di una rettifica legislativa finalizzata al ripristino di una presunta reciprocità, come è stato detto da qualcuno, ma è un ribaltamento in punta di diritto, di principio e di buonsenso. E sarei veramente curioso di capire quale complesso ragionamento scientifico abbia condotto a questo risultato. in tale modo si svilisce quel percorso storico-politico a cui facevo riferimento, ma perché, con un colpo di spazzola, si superano anche i principi costituzionali che all'epoca ne hanno decretato la legittimità. Come è stato già evidenziato, l'istruttoria legislativa del 2001 venne arricchita anche dal contributo del parere di autorevoli costituzionalisti che, riletti oggi, sono di un'attualità disarmante, e che si orientavano tutti nella medesima direzione. Essendoci state precedenti revisioni costituzionali con le quali fu istituita la circoscrizione estero, la limitazione dell'elettorato passivo non solo non è in contrasto con i principi di uguaglianza e di libertà, ma costituisce la conseguenza logica, necessaria, del dettato costituzionale. Lungi da me svolgere un approfondimento dell'analisi costituzionale, non essendo questa la sede più congeniale, ma non posso esimermi dal citare alcuni passaggi di pareri: a titolo di esempio il parere del professor Baldassarre (richiamato in più occasioni anche dal mio collega Micheloni), quale evidenziava come la *ratio* della norma fosse garantire che gli italiani residenti all'estero siano rappresentati da persone che condividono la loro stessa condizione e la loro stessa esperienza, evitando - e sottolineo questo punto con enfasi - che siano colonizzati da candidati paracadutati dal territorio nazionale. Inoltre, nel parere si evidenziava come la norma diretta a realizzare l'interesse costituzionale relativo alla genuina espressione della liberta di voto e all'effettivo ed eguale esercizio della medesima libertà. A tale parere si aggiunge tra gli altri quello del professor Fusaro che, tra le altre cose, evidenziava quanto fosse azzardato discutere della ragionevolezza di una norma che vuole introdurre un elemento di garanzia del nesso di collegamento territoriale tra elettori ed eletti della particolarissima circoscrizione estero. E sottolineava ulteriormente il rischio di candidature ad effetto che potrebbero svuotare la ragione stessa dell'istituzione della circoscrizione estero, portando all'elezione di personalità di alcun legame con i propri rappresentati e difficilmente in grado di garantire quello specifico tipo di rapporto rappresentativo che la modificazione costituzionale ha inteso rendere possibile. Vale la pena dire, quindi, che il combinato disposto di illegittimità costituzionale ed incoerenza storico-politica fa di questo disegno di legge un precedente pericoloso. Queste sono le premesse, ma andiamo nello specifico. Le modifiche apportate all'articolo 8 della cosiddetta legge Tremaglia sono una breccia nel sistema, e lo dico con cognizione di causa. Possiamo facilmente immaginare che dinamiche avranno le ipotetiche candidature colonizzanti: penso ai referenti di gruppi malavitosi attivi all'estero, già operativi sul fronte della cooptazione di voti, attraverso le comunità regionali che stanno già vivendo questa pressione, passando per pseudo-imprenditori conniventi e operanti ai limiti della liceità, che detengono gli strumenti economici per sostenere le sostanziose campagne elettorali oltre confine. Ciò senza trascurare

pari allo zero. Come si potrebbe definire questa operazione, se non una delegittimazione radicale del voto di quasi 4 milioni di cittadini nel mondo? La volontà di svilimento del diritto di rappresentanza dei cittadini residenti oltre confini non comincia certo oggi. La mancanza di riscontri, il ridimensionamento dei fondi, la razionalizzazione della rete consolare tutti segnali sicuramente chiari, che assumono un significato forse più evidente e risolutivo con questo ultimo affondo legislativo, che si configura come l'atto ultimo dello smantellamento della ripartizione estero e della sua ragion d'essere. La modifica in questo disegno di legge è stata giustificata dall'urgenza di ristabilire la reciprocità tra cittadini in Italia e quelli residenti all'estero, ma un'interpretazione estensiva di questa stessa reciprocità imporrebbe qualcosa in più da parte di coloro che si sono battuti per questo principio. Infatti, verrebbe da chiedersi: in nome di questa presunta reciprocità avevate l'obiettivo di intervenire sulla disciplina, ma perché non ve ne prendete tutte le responsabilità? Avete lasciato alla disciplina originaria le cose più comode per qualcuno, come l'onere dell'opzione per i cittadini residenti all'estero e la sussistenza di un sistema elettorale differente basato sul proporzionale di preferenza.

Avete preferito intraprendere la strada più complicata e indifendibile per fare passare una modifica che ha soltanto motivazioni di bassa politica, trascurando gli esiti che tutto questo avrà in termini di coerenza costituzionale, credibilità e rispetto storico. Trasformare una storica conquista di democrazia in un contenitore vuoto attraverso cui veicolare una nuova gabella politica è un'impresa ragguardevole. Di tutto questo vi dovete assumere le vostre responsabilità. Resta l'amarezza per non aver fatto saltare questa incursione alla Camera, in una legge necessaria, ma insostenibile, per quanto riguarda la circoscrizione estero. Sono certo, facendomene garante, che la legittimità di quanto introdotto verrà opportunamente contraddetta nelle opportune e adeguate sedi. È presente in tribuna una delegazione di ELSA (Associazione europea studenti in legge), sezione di Catania, che segue i nostri lavori e che salutiamo.

sento il bisogno di testimoniare il fatto che non sono d'accordo con le scelte fatte né nel metodo né nel merito. Noi passeremo ai libri di storia. Questa giornata verrà ricordata sui manuali e si dirà che è stata la prima volta che, su un disegno di legge elettorale così delicato e importante per il rapporto tra cittadini e istituzioni, il Governo ha posto la fiducia due volte, alla Camera e al Senato. e al Senato. Voglio dire che su questo non ero d'accordo e non sono d'accordo. Non sono d'accordo nemmeno su molti dei contenuti di questa legge, che viene fatta in un modo proditorio a pochi mesi dalle elezioni. Da questo punto di vista, mi chiedo quanto di europeo ci sia in questo comportamento, quanto dell'appartenenza all'Europa portiamo in in questa Assemblea dopo che l'Europa ha detto esplicitamente che non è il caso di legiferare a pochi mesi dalle elezioni in materia elettorale.

Uno dei problemi più grandi che abbiamo è ristabilire una fiducia, un legame tra cittadini e istituzioni, tra il popolo italiano e questo Parlamento, molte volte bistrattato, e questo ramo del Parlamento, che si è provato anche a chiudere in modo così poco dignitoso.

partecipazione. Uno degli elementi importanti nella discussione di una legge elettorale, in una fase come questa, è in che modo i cittadini possono partecipare alla selezione

e che permettevano una certa selezione con una partecipazione abbastanza ampia. Un altro modo è la possibilità di trovare anche sistemi nuovi per selezionare i i candidati delle liste, e secondo me sarebbe stato importante per dare valore al modo in cui i cittadini si organizzano per partecipare alla vita del Paese.

se questa cosa non succede, viene rilevata ma non sanzionata. Non c'è nulla, non c'è nessuna cancellazione delle candidature eccedenti di un sesso o dell'altro, e secondo me questo è un elemento di sciatteria, da una parte, ma è anche una scelta politica precisa dall'altra, signor Presidente. Noi siamo un Paese che anche in questo modo segna il suo elemento di arretratezza nelle questioni di rappresentanza di genere e di parità. A livello europeo la parità della rappresentanza viene assunta da molti movimenti di donne, ma anche da molti Governi, come

di molti movimenti, ma anche di molti Governi, c'è stata un'elaborazione costante su cosa significa la partecipazione alle assemblee elettive delle donne

onorevoli colleghi, in questa legislatura il tema della legge elettorale è stato affrontato come mai nel passato, anche per il verificarsi di fatti nuovi come l'intervento in questa materia da parte della Corte costituzionale. In particolare, le modalità proprie di azione della Corte costituzionale ne hanno in verità dimostrato anche i pesanti limiti. Infatti, in mancanza del provvedimento che ci apprestiamo a varare, le sentenze restituiscono un impianto elettorale di dubbia applicabilità. Siamo quindi in un'Assemblea preparata su questo tema e, secondo la mia opinione, ciò dovrebbe consentire un confronto carico di consapevolezza. Essendo a disposizione di tutti riflessioni autorevoli e, a mio avviso centrate, svolte nelle audizioni in Commissione (come quella, tra le altre, di Carlo Fusaro), mi limiterò ad alcune sottolineature per dare il senso delle scelte di fondo che costituiscono la linea di coerenza di questo disegno di legge elettorale. La legge elettorale deve trasformare il voto di circa 47 milioni di italiani in 630 deputati e 315 senatori. In questo sarebbe auspicabile che ci fossero possibilità per il formarsi di maggioranze politicamente omogenee per garantire un Governo stabile nel Paese. In altre parole, la legge elettorale è uno strumento che dà equilibrio tra rappresentanza e governabilità. Dopo i *referendum* del 1991 e del 1993 inizia il percorso in questo senso e si consolida la convinzione che il cittadino dovrebbe votare conoscendo prima le compagini che si propongono di governare, eliminando anche le preferenze che hanno sempre portato al prevalere di aspetti patologici. Prima di allora il cittadino votava soddisfatto il partito che rispondeva al 100 per cento alle proprie aspettative, pensando che poi avrebbe realizzato il programma elettorale proposto, salvo poi vedere che il giorno dopo le elezioni quello stesso partito andava a sedersi con altri a concordare cose diverse da quelle promesse. Bene, ora il contesto nel quale ci troviamo è quello del dopo 4 dicembre 2016, una data spartiacque. Sapevamo che lo sarebbe stata in ogni caso, ma nel caso che si è verificato lo è in un senso che riguarda essenzialmente la legge elettorale. Non avendo modificato il sistema parlamentare che avrebbe dato un profilo pienamente maggioritario al sistema, quegli obiettivi che ho appena enunciato vanno ora perseguiti differentemente attraverso la legge elettorale. Si potrebbe dire che, vista la situazione, la scelta più semplice sarebbe stata tornare alla cosiddetta legge Mattarella. Noi l'abbiamo sempre dichiarato e l'abbiamo anche riproposta a destra e soprattutto a sinistra. Chiedete all'onorevole Giachetti come è andato il confronto sulla cosiddetta legge Mattarella in questa legislatura. Non c'erano i voti per approvare la legge Mattarella e non ce ne erano neppure per altre leggi maggioritarie possibili. Dopo un duro contrasto politico, che ha visto soccombere l'idea di una polarizzazione sui partiti principali, ma anche il concetto di governabilità, il sistema politico ha inevitabilmente virato sul proporzionale e sulla logica di coalizione, ricercando un accordo su questo sistema. Questa, la legge Rosato, è una legge semplice. Si votano le coalizioni e si votano i partiti che le compongono, i quali si assumono la responsabilità riguardo alla credibilità della compagine e delle persone che la rappresentano, senza voto di preferenza, come da venticinque anni a questa parte. Un sistema prevalentemente proporzionale, con una parte maggioritaria con collegi uninominali: la coalizione dei partiti è chiaramente riconoscibile nella scheda ed è chiaramente collegata al candidato uninominale. Se qualcuno non vuole fare coalizioni, non ci sarà alcun dubbio riguardo al partito sul quale verrà riversato il solo voto al candidato uninominale. Su questa legge c'è una larga maggioranza - il tabellone illuminato per la controprova del voto sulle pregiudiziali lo ha mostrato chiaramente che va oltre quella di Governo; coloro che la sostengono hanno trovato un punto medio su cui convergere, rinunciando a molto di ciò che avrebbero preferito. Altro di più preferibile, direi ben altro, non ha i voti per essere approvato, ma ciò che stiamo per votare migliora responsabilmente il quadro incoerente restituito dalle sentenze della Corte. Altrettanto incoerenti sono le critiche sollevate da chi si oppone. Da tutte le singole critiche sentite in questi giorni non esce una legge alternativa che stia insieme e tanto meno che riesca ad essere approvata: il premio di maggioranza di Fratelli d'Italia, le soglie alte di MDP, tutti i sistemi e il loro contrario proposti dal Movimento 5 Stelle, come dimostrano gli emendamenti presentati Con questa legge rispondiamo seriamente alle indicazioni della Corte costituzionale e alle attese del Capo dello Stato. E, proprio perché è una legge semplice, i cittadini sapranno utilizzarla per dare un'indicazione chiara sul futuro del Paese.

Signor Presidente, il disegno di legge elettorale mi scaraventa in un paradosso. Da un lato condivido tutto e dall'altro non condivido niente. Siamo alla fine della legislatura e c'è in Aula una proposta per superare il vigente Consultellum, che sarebbe la peggiore soluzione, non solo per le sue gravi anomalie, ma per la definitiva delegittimazione del Parlamento. Se fosse solo questo, non potrei che votare a favore. Ma non riesco a non domandarmi: come siamo arrivati fin qui? E soprattutto, con quali forzature istituzionali? E quali inganni contengono queste norme? La legislatura si chiude come si era aperta, con strappi inusitati allo stile repubblicano. La legge elettorale si doveva approvare subito dopo la sentenza della Corte sul Porcellum. Invece, in contrasto con il buonsenso, si affidò l'arduo compito di riscrivere la Costituzione a un Parlamento eletto con legge incostituzionale. È stato l'inizio di tutti gli errori successivi e ne portano la responsabilità in tanti, sia chi comanda adesso nei partiti, sia chi allora ne era a capo. Oggi non si può accettare il voto di fiducia sulla legge elettorale. Non si invochi il caso della legge truffa, perché allora il Presidente del Senato respinse la richiesta di voto di fiducia e poi di dimise dalla carica. Era un vecchio liberale, come se ne trovano pochi oggi in Italia. L'altro precedente è l'Italicum, che meritava solo l'oblio, almeno per un senso di pudore. Sono caduti tutti i freni inibitori: anche la mozione contro la Banca d'Italia conferma che perfino i propositi più sconvenienti possono essere messi ai voti. Ormai si può fare tutto, se è funzionale a uno scopo. Il ceto politico non è più capace di darsi liberamente dei limiti, di fermarsi prima di apparire sguaiato, di evitare ciò che è inopportuno, anche se non è vietato. Le pulsioni politiche perdono ogni riguardo, svestendosi delle forme istituzionali. Se manca il senso del pudore si rischia di perdere anche il dovere della responsabilità. Il limite della politica è l'essenza di ogni Costituzione. Non si era mai arrivati a utilizzare il voto di fiducia in accordo con una parte dell'opposizione per ratificare una intesa raggiunta dai capi partito fuori dal Parlamento, senza una adeguata istruttoria nei Gruppi e nelle Commissioni parlamentari. Non si era mai arrivati a utilizzare il voto di fiducia per una banale questione di agenda extraparlamentare, per l'ossessione di concludere prima delle elezioni siciliane. Il voto di fiducia oggi, qui, non delimita il confine tra maggioranza e minoranza ma mostra la frattura tra i parlamentari, chiamati solo a ratificare, e i capipartito di maggioranza e minoranza, che decidono da soli. Questi hanno anche il vezzo di inserire nella legge elettorale l'inedito *status* di capopartito, fino a insidiare le prerogative del Quirinale sull'incarico di Governo. Eppure, dovrebbero essere *leader* forti. Così si sono raccontati in questi anni. Sembravano capaci di grandi imprese, protesi verso plebisciti popolari. Eppure, non riescono neppure a convincere i propri parlamentari. Ricorrono a vincoli di legge perché hanno desertificato la democrazia interna dei loro partiti. Oggi mi si chiede disciplina. Come senatore ho potuto seguire solo sui giornali il dibattito sulla legge elettorale. Il Gruppo a cui appartengo, ma credo valga anche per qualcun altro, non è mai stato riunito se non per ratificare l'esito finale; in altri tempi, i senatori sarebbero stati coinvolti in sede politica anche se la legge fosse stata incardinata alla Camera. Per la prima volta in epoca repubblicana il Senato non è messo in grado di discutere ed emendare una legge elettorale secondo procedure normali. Se le cose seguiteranno così, si finirà per dare ragione a chi propose di delegare l'attività legislativa alla riunione dei Capigruppo. Con la stessa logica fu approvato il Porcellum per affidare ai capipartito la nomina dei parlamentari, sottraendo di fatto la scelta agli elettori. Eppure - mi rivolgo ai senatori della destra - devo riconoscere, non senza sofferenza, che quella di Berlusconi fu un'invenzione lungimirante, perché tracciò una via che nessun'altra forza politica seppe abbandonare. Tutti i disegni di legge elettorali arrivati all'esame dell'Assemblea in questa legislatura, anche il finto modello tedesco condiviso dal Movimento 5 Stelle, hanno avuto un unico punto fermo: l'indebolimento del potere degli elettori nella selezione degli eletti. Quella innovazione, tanto lungimirante negli effetti quanto sciagurata nei contenuti, coglieva una tendenza strutturale della politica dei tempi nostri. Il *leader* mediatico cerca una legittimazione diretta con il proprio popolo e non può tollerare l'esistenza di un altro canale di legittimazione diretta tra eletto ed elettore. L'uomo solo al comando ha bisogno di un Parlamento debole e screditato. Viene dall'alto, non dal basso, la corrosione populistica delle istituzioni. Il Porcellum è l'evento politico più importante della politica italiana di questo inizio secolo. Ha spezzato la relazione eletti-elettori che si alimentava, pur con tanti limiti, nei collegi del Mattarellum. Da quel momento si è accentuata la separazione della classe politica dal Paese reale ed è iniziata la polemica sulla casta che ha portato poi a destrutturare il breve bipolarismo. Sarebbe il tempo per una svolta, e invece si prosegue nella vecchia strada. Di più, gli elettori sono ingannati tre volte. II primo inganno è nell'incatenamento del voto tra uninominale e proporzionale. Sostenendo il candidato di collegio, l'elettore è costretto a votare alcuni partiti senza averli scelti. Il secondo inganno è nella coalizione, che serve solo a raccogliere voti ma non diventerà mai un'alleanza di Governo. Si promuovono tante liste di ambito locale o di argomenti particolaristici che andranno a rafforzare i consensi del *leader*, anche senza una proposta programmatica di coalizione. L'esito sarà un Parlamento più frammentato e più ingovernabile. Il terzo inganno è nel votare senza poter conoscere tutti gli effetti del voto. Le norme sono tanto confuse da prevedere perfino che l'Ufficio elettorale possa dotarsi di esperti per interpretarle. Ma le regole elettorali dovrebbero essere facilmente comprensibili per i cittadini. Non posso approvare questa legge che conserva la politica italiana nella palude dell'ultimo decennio. Per uscirne bisognava cancellare per sempre la logica del Porcellum, delle liste bloccate e anche delle preferenze. Si doveva ricostruire un rapporto diretto tra eletti ed elettori, collegando ogni deputato a un collegio piccolo come un quartiere di città o una unione di Comuni. Un'Assemblea di oltre 600 deputati legati a piccoli collegi sarebbe una Camera stimata dai cittadini, sovrana nella politica nazionale, autorevole tra le istituzioni europee. Sarebbe l'*incipit* di una nuova stagione della democrazia italiana.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, diciamo no, fieramente no alla nuova legge elettorale, il Rosatellum, l'Imbroglioncellum o il Verdinellum, che dir si voglia. Il no di Articolo 1 è un no indignato, anzitutto nel metodo utilizzato: una legge elettorale approvata a cinque mesi dalle elezioni politiche, in quella zona Cesarini in cui l'Europa stessa ci dice che non bisogna procedere al cambiamento delle regole del gioco, e per di più imponendo in prima lettura la fiducia sia alla Camera sia al Senato, realizzando una violenza istituzionale verso il Parlamento senza precedenti nell'intera storia d'Italia. Vi assicuro che questo passaggio finirà nei manuali di storia. State scrivendo una pagina di cultura costituzionale di cui, presto o tardi, vi dovrete vergognare. State tradendo quei principi che sono nella carta dei valori del Partito Democratico e nella storia della sinistra italiana. Ci sarà pure un motivo se dal 1861 a oggi nessun Governo - liberale, fascista, o democratico - sotto la monarchia o sotto la Repubblica ha mai osato imporre la fiducia in entrambi i rami del Parlamento. Tra l'altro, state creando un pericoloso precedente che si configura come la messa in pratica di una vera e propria dittatura della maggioranza: dopo di voi qualunque Governo si sentirà autorizzato a mettere la fiducia su qualsiasi legge elettorale a pochi mesi dalle elezioni, facendo coincidere la maggioranza di Governo con la futura ma prossima coalizione politica. E se la legge avesse anche degli elementi di incostituzionalità, poco male perché il giudizio della Suprema Corte interverrebbe dopo - anche molti anni dopo - e intanto il Parlamento si sarà formato in forza di quella prepotenza, a immagine e somiglianza degli interessi di una sola parte. Proprio questo è quello che sta avvenendo nelle ultime ore. Si è perso tempo - come è già avvenuto con l'infausta esperienza dell'Italicum per creare le condizioni di emergenza che impongono la fretta e, dunque, la fiducia. Tre sono i limiti strutturali, a giudizio di Articolo 1, di questa legge, alcuni dei quali hanno un chiaro profilo di incostituzionalità che contribuisce ad aumentare il discredito dell'istituzione parlamentare davanti all'opinione pubblica, perché dopo il Porcellum e l'Italicum non c'è due senza tre. limite riguarda la permanenza di un Parlamento a maggioranza di nominati, scelti dal capo di turno, con una grave lesione del principio di rappresentanza. Errare è umano, ma perseverare è diabolico. È dal 2006 che i parlamentari italiani sono cooptati e ciò ha contribuito ad aumentare il fossato tra cittadini e Parlamento, gettando benzina sul fuoco dell'antipolitica e delle forze antisistema che - non a caso - proprio negli ultimi dodici anni sono prosperate. La nomina del parlamentare espropria il cittadino di un supremo diritto di scelta, trasformandolo in un semplice potere di ratifica.

che amplifica il trasformismo e rimane tutta interna al Palazzo, al ceto politico, che a questo punto viene giustamente considerato una casta separata e chiusa nei suoi privilegi, senza rappresentanza. Il secondo limite riguarda la pesca a strascico del voto: una sorta di supermercato elettorale con cui paghi uno e prendi tre. Qui sussiste - a mio giudizio -un possibile profilo di incostituzionalità del Rosatellum: il voto del cittadino si trasforma in una pallina di flipper, in cui le intenzioni e le volontà iniziali dell'elettore rischiano di avere conseguenze pratiche così distanti ed evanescenti da essere tradite. Il terzo limite punto riguarda l'assenza di un incentivo alla governabilità e la chiara scelta, con soglie minime e incoerenti - dall'uno per cento delle liste civetta al tre di frammentare il più possibile il prossimo Parlamento, per ulteriormente svilirlo e indebolirlo; un veleno funzionale - di questo si tratta - ad assicurare una governabilità fragile e mediocre; un governicchio di minoranza tra Renzi e Berlusconi, che non potrà essere all'altezza dei problemi dell'Italia, ma solo a garanzia degli interessi di fazione di due gruppi di potere. Osservate un attimo, colleghi: nel giro di due anni Renzi è passato da tre diverse fasi che testimoniano chiaramente come egli abbia non un disegno per l'Italia e per la qualità della sua democrazia, ma soltanto una spasmodica volontà di resistere al potere, nonostante le numerose smentite del voto degli italiani, prima e dopo il 4 dicembre. In una prima fase il mantra era quello di sapere la sera stessa delle elezioni chi fosse il vincitore, quando Renzi e il PD pensavano di essere loro. In una seconda fase si è fatto di tutto per cambiare l'Italicum - ovviamente votando sì al *referendum* - ma eliminando il ballottaggio, quando si è capito che quella fatidica sera i vincitori avrebbero potuto essere gli altri, ossia i 5 Stelle o la destra. Ora, invece, si vuole una legge che non dia nessun vincitore, così da rendere inevitabile l'abbraccio con Berlusconi e Verdini. Per questa ragione, il Rosatellum è un atto di forza e di arroganza, Per la prima volta, colleghi, le larghe intese sono non una conseguenza - amara e obbligata - del risultato elettorale, ma una scelta preventiva, cercata e voluta addirittura in sede di elaborazione della stessa legge. Qui sta il grande inganno del Rosatellum, che è la storia di un grande tramonto del berlusconismo e del renzismo insieme, che gli italiani sapranno giudicare e punire alle prossime elezioni.

Partita e già quasi data per morta, la XVII legislatura sembrava all'inizio dovesse durare appena il tempo necessario a convocare nuove elezioni, travolta da un risultato elettorale che si è rivelato essere un vero e proprio terremoto per il tradizionale sistema bipolare. Poi, però, c'è stato il Governo Letta che doveva durare fino alla fine del semestre italiano, e invece è arrivato Renzi e la legislatura ha avuto l'aspirazione di diventare costituente. Sappiamo, tuttavia, come è andato a finire il *referendum* e sappiamo come sono andate a

E così adesso ci troviamo di fronte agli ultimi atti di una legislatura che non ha saputo dare una soluzione al nuovo assetto tripolare del sistema partitico italiano, e che si accontenta di limitare i danni che, dal punto di vista della legislazione elettorale, ha prodotto in questi anni: da legislatura di transizione a legislatura di transizione, si potrebbe dire; una transizione verso un'ipotetica Terza Repubblica che ancora una volta però nascerebbe senza una vera riforma costituzionale, ma solo tramite la legislazione elettorale e un terremoto nell'offerta politica; una Terza Repubblica che, tra l'altro, rischia di assomigliare molto alla Prima. La legge elettorale che stiamo discutendo sembra il frutto dell'ultima fase della legislatura, seguita alla bocciatura della riforma costituzionale e alla sentenza della Corte costituzionale sull'Italicum. D'altra parte, se in questo Parlamento ci fosse maggiore senso di responsabilità e non ci fosse una forza politica che confonde la normale dialettica parlamentare e il compromesso politico con l'inciucio, avremmo potuto trovare accordi più ampi, e forse migliori, lavorare in tempi più ragionevoli, e non ridurci ad approvare una nuova legge a pochi mesi dalle urne. Quando si cambiano le regole a pochi mesi dal voto si è già sbagliato, qualunque sia l'esito finale della discussione. Si ricordino al riguardo le raccomandazioni della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa in materia elettorale: non si dovrebbe modificare la legge elettorale a un anno, e quindi, a maggior ragione, a pochi mesi dalle successive elezioni. Quando questo accade, inevitabilmente le forze politiche finiscono per studiarla sondaggi alla mano. Ed è innegabile che questa proposta di legge abbia al suo interno optato per alcune scelte tecniche volte ad avvantaggiare chi questa legge infatti sostiene e vuole approvare. La legge in discussione, per entrare nel merito, non fa più danni di quelli che avrebbero fatto altri sistemi elettorali. In un sistema così tripolare, dati gli attuali dati e sondaggi, il Rosatellum non darà una maggioranza di Governo che corrisponderà a uno degli schieramenti che si presenteranno agli elettori. Ma, con tutte le simulazioni fatte in questi mesi, nessuna delle proposte fatte dava un differente esito. Cambia poco, in termini di «Governo scelto il giorno delle elezioni», tra questa legge e le opzioni avanzate nei mesi scorsi. Siamo passati da da un sistema che dava la certezza di avere una maggioranza alla Camera dei deputati, a qualsiasi costo di disproporzionalità (l'Italicum), a una legge che ci dà la certezza di non avere maggioranze in entrambi i rami del Parlamento. Si guardi a tal proposito la griglia proposta da D'Alimonte sul sito «cise.luiss.it» per avere immediatamente un'idea di quanto sia difficile avere una maggioranza parlamentare senza un consenso elettorale vicino al 50 soglia che ragionevolmente non sarà raggiunta né dal centrodestra, né dal centrosinistra, né, tantomeno, da un partito che non è di centro, di destra e di sinistra. Sarebbe forse stato opportuno mantenere un piccolo premio di governabilità, magari anche solo alla Camera, giusto per dare agli elettori un potere di indirizzo nella formazione dei Governi *post* elettorali, ma si è deciso diversamente. Possiamo comunque dire che tanto abbiamo ascoltato elogi alla democrazia dell'alternanza, sulla necessità di superare la stagione delle larghe intese - idea democratica per la quale era necessario a qualunque costo approvare l'Italicum che appare oggi un gran salto concettuale discutere di una legge che in alcune sue scelte risulta rimandare chiaramente a una logica consensuale e di Governi di coalizione *post* elettorale. Basti pensare alla prudenza con la quale si parla di coalizioni: solo un terzo dei seggi, senza programma comune, senza l'indicazione di un *leader* politico di coalizione. Appaiano obiettivamente dei cartelli elettorali volti ad ottenere più seggi. Per carità, se vogliamo sono scelte oneste e coerenti con quello che, con ogni probabilità, sarà necessario fare dopo le elezioni: ossia sciogliere le coalizioni elettorali per dare un Governo a questo Paese. E allora la scelta del legame debole tra le forze coalizzate prima del voto è onestà nei confronti dei cittadini. Ma viene il dubbio che le coalizioni così pensate passino alla storia come un retaggio di una stagione finita, a meno che il Rosatellum - come credo - in realtà, avrà breve vita e, nel momento stesso che il sistema partitico si sentirà sufficientemente al sicuro da ulteriori terremoti, si tornerà ad aumentare l'impronta maggioritaria al fine di facilitare la tradizionale alternanza tra centrosinistra e centrodestra. Vedremo. Noi oggi ci troviamo senza alternative. Le leggi della Consulta andrebbero comunque armonizzate e sarebbe comunque sempre questo Parlamento chiamato a farlo, manifestando le stesse volontà politiche che hanno condotto al disegno di legge in discussione oggi. Per cui, anche chi ritiene che si doveva partire dalle leggi della Consulta dovrebbe ammettere che il risultato finale non sarebbe stato molto distante da quanto stiamo votando. Il Rosatellum può forse essere inteso, da un certo punto di vista, come l'armonizzazione delle due leggi uscite dalle sentenze della Corte costituzionale: avevamo un sistema sostanzialmente proporzionale con potenziali correttivi maggioritari alla Camera dei deputati - il premio era difficile da ottenere, ma era presente - e correttivi maggioritari effettivi al Senato,

C'erano le coalizioni al Senato e non alla Camera e con il Rosatellum abbiamo delle coalizioni che - come abbiamo già detto - sono piuttosto deboli. Abbiamo una soglia ragionevole al tre per cento e, per il resto, ci troviamo di fronte a un impianto proporzionale con correttivi, esattamente com'è l'impianto del sistema elettorale fuoriuscito dalle sentenze, con il vantaggio non indifferente di avere un sistema pressoché uguale tra Camera dei deputati e Senato, come da tutti richiesto. Per quel che riguarda la rappresentanza di genere, essa è stata armonizzata, ma forse in maniera *sui generis*, come già altri parlamentari hanno detto. Il Movimento 5 Stelle grida allo scandalo, ma di fatto lo fa perché ritiene che il disegno di legge al nostro esame possa danneggiarlo. In realtà anche questo è vero solo in parte: dipenderà molto dal comportamento strategico dell'elettore, che al momento è difficile da prevedere. Rimane sul tavolo la questione delle preferenze, un tema che negli ultimi decenni ha conosciuto senza dubbio alterne fortune: da anomalia, da male profondo della politica italiana - tanto da indire un *referendum* nel 1991 - a strumento a strumento principe per la difesa del potere di scelta dei cittadini. Sulle preferenze si possono avere opinioni differenti, ma sicuramente il listino corto bloccato non è incostituzionale e può anche essere interpretato come una scelta coerente in un sistema misto, dove la scelta del candidato vicino al territorio dell'elettore viene offerta tramite i collegi uninominali: scelta giustificata, legittima e coerente, quindi, se non fosse che la legge non consente il voto disgiunto e l'elettore si trova di fronte a un pacchetto da scegliere, che vincola la scelta alla lista a un candidato predeterminato nel collegio uninominale. Obiettivamente questo è il punto più contradditorio della legge e andrebbe modificato, ma ovviamente non si può fare, dal momento che è stata fiducia. Risulta davvero difficile da giustificare la scelta di negare il voto disgiunto ai cittadini: si perde la *ratio* di avere un sistema misto e i collegi uninominali, anche se - pure nel caso del voto disgiunto come in quello delle preferenze - non si dovrebbero esacerbare gli animi per strumenti che poi, laddove sono consentiti, non vengono certo utilizzati dalla maggior parte dei cittadini. Un esempio su tutti è la virtuosa Germania, in cui, mediamente, vota in modo disgiunto non più del 20 per cento dei votanti. Nell'Italia delle preferenze, il cittadino comune vota generalmente il simbolo, senza indicare alcuna preferenza, anche quando era

d'Italia. In definitiva ci troviamo a votare una legge che non risolverà i problemi di governabilità o, quantomeno, non nel senso che oramai si tende a dare a questa parola - ossia non avremo un vincitore chiaro il giorno delle elezioni, con una propria forte maggioranza che non dovrebbe incorrere in vizi di costituzionalità e armonizzare le leggi in vigore per le elezioni delle due Camere. Di questi tempi possiamo dire che non è poco.

avrei voluto parlare in quest'Aula del merito delle modifiche al sistema di elezione della Camera e del Senato della Repubblica. Avrei voluto parlare delle modifiche che portano alla determinazione di collegi elettorali uninominali e plurinominali di tipo ben diverso da quelli

Volevo esplicitare, in quest'Aula, le conseguenze per il Paese di un sistema elettorale misto, che non offre all'elettore la possibilità di esprimere un voto disgiunto tra collegio uninominale e lista. Noi non crediamo affatto che possa esserci una relazione tra queste liste di coalizione e la migliore governabilità del Paese. Ma avete fatto ricorso anche in questa Camera allo strumento ignobile della fiducia, uno strumento applicato in un'Aula parlamentare dopo che è già stato applicato nell'altra. Ed è fin troppo evidente che non si è voluto assicurare una fedele rappresentazione della volontà del votante e l'interesse prioritario è quello di poter liberamente utilizzare i voti espressi nei singoli collegi con una libera distribuzione a livello nazionale. Quanto ai contenuti della legge elettorale, vi sono molti elementi di dubbia legittimità costituzionale ed è sicuramente grave impegnarsi, solo a pochi mesi dal voto, per definire un testo che si può dire non voluto da una larga maggioranza dei partiti, ma piuttosto gradito alla maggioranza dei partiti che trovano in esso la maggior garanzia di assicurarsi posti per i loro prediletti e di mantenere in piedi un sistema politico-sociale costruito da più di vent'anni, che sta manifestando il peggio in questa ultima legislatura. Rinuncio a proseguire in una discussione nel merito, perché voi non ci avete garantito la possibilità di discutere e di emendare nel merito, di correggere le storture e di avanzare le proposte migliorative. Rinuncio a svolgere il mio intervento, consapevole, purtroppo, che per questo ennesimo sopruso normativo realizzato in quest'Aula non ci sarà il vaglio del voto referendario che ha già bloccato il 4 dicembre lo scellerato tentativo di trasformare il Senato in un'inutile Camera delle Regioni, fingendo un risparmio che non ci sarebbe mai stato. Ma la sovranità popolare potrà ancora manifestare il suo volere, soprattutto se gli astensionisti, che sono sempre stati la vera maggioranza del Paese, torneranno a votare con il disgusto per queste consuetudini

l'ha manifestata arrivando a lanciare un appello poche ore fa, nonostante voi continuiate a negarla e a contenerla, evitando che i nostri interventi vengano ascoltati dai giovani e dai giornalisti, come avete fatto con il cambiamento degli interventi previsti già dal calendario, modificato con continui inserimenti senza logica. Ripeto che la consapevolezza della cittadinanza c'è e ne sta prendendo atto anche il signor Renzi, che gira in *tour* con un treno, a imitazione del Movimento 5 Stelle. Ma l'originale è sempre meglio delle imitazioni farlocche.

la discussione delle ultime ore e, più in generale, la modalità con la quale la maggioranza e il Governo hanno deciso di fare la legge elettorale il triste, e forse inevitabile, epitaffio di questa legislatura. triste epitaffio inaccettabile nel metodo - come è stato ricordato da diversi colleghi - e non devo aggiungere altre parole su come questa scelta segni un precedente

Come vi ho detto varie volte in quest'Aula e vi ripeto anche stasera, anche se siamo rimasti in pochi - forse neanche la discussione interessa più di tanto quest'Aula del Senato - state davvero scherzando con il fuoco. fuoco. Il Paese è segnato così profondamente dalla crisi sociale ed economica; è un Paese segnato dalla crisi morale; un Paese che non riconosce più le sue classi dirigenti e vede una parte sempre più grande dei cittadini italiani non andare nemmeno più a votare o votare partiti e movimenti che hanno programmi politici di grande contestazione e di grande rottura rispetto a quanto è successo negli ultimi anni.

Avreste avuto l'obbligo politico, forse finanche morale, di capire che, dinanzi a un *vulnus* così serio della democrazia italiana, dovevate mettere in campo tutti gli strumenti atti a colmarlo o almeno a cambiare la tendenza che, pure drammaticamente, si è dimostrata e costruita in questi anni. Invece, ancora una volta scegliete una modalità - è anche un merito della riforma - che questo *vulnus* accentuerà ancora di più. Non ci sarà cittadino del nostro territorio che non penserà nelle prossime ore che, ancora una volta, questo Parlamento appare distante anni luce da un Paese reale da un Paese reale che non capisce più la lingua che si parla qui dentro e che vi ha anche mandato a dire che non capiva più niente delle vostre scelte e della vostra politica. Avevate già sbagliato tutto, colleghi della maggioranza di Governo, quando avevate pensato di imporre la riforma costituzionale a colpi di maggioranza: ve l'avevamo detto. Eravamo in pochi quando cominciammo la battaglia contro la vostra riforma costituzionale, ma man mano, giorno dopo giorno e mese dopo mese, siamo cresciuti fino a diventare maggioranza schiacciante di questo Paese. La vicenda che si è consumata in quei giorni

Si prende coscienza del fatto che, quando uno schiaffone è così potente, forse il popolo italiano ti sta chiedendo e indicando la possibile via di uscita dalla crisi democratica che si è consumata in questi anni. La soluzione della crisi democratica è un gioco di parole, ma è l'unica possibile verità: è più democrazia. Non c'è altra soluzione rispetto a questo.

una proposta di legge che abbia altre caratteristiche rispetto all'idea di fondo solennemente bocciata dal popolo italiano.

verso questo Senato della Repubblica. In quella bocciatura c'era, invece, l'idea profonda che dinanzi alla crisi bisognasse rispondere invertendo radicalmente la tendenza

Come fate a non vedere che giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno diminuisce in maniera drammatica la percentuale dei cittadini che vanno a votare? Come fate a non vederlo? Questa legge elettorale,

Come fate a non vedere che queste scelte non faranno altro che favorire ancora di più quei movimenti e forze politiche che hanno fatto dell'anti politica, della critica ai partiti e al sistema

di chi ha costruito attorno alla critica al vostro sistema politico la sua principale ragione di consenso? Come si fa a non vedere quanto sta accadendo? Come si fa a non vedere che questa miscela

alla cittadinanza di questo Paese e di rimettere in piedi alcuni elementi minimi di democrazia, di partecipazione, di coinvolgimento popolare. Non avvertite questa distanza siderale?

sacrifici e che in questo Paese è stato il grande caposaldo attorno al quale si è costruita la democrazia italiana? Come fate a non vedere quello che sta accadendo? Come fate a essere ciechi dinanzi a segnali così evidenti? Insomma, attraversano tutta l'Europa. Cosa deve più accadere anche nel resto del continente europeo? Vedete cosa sta succedendo ai partiti politici dei principali gruppi che hanno segnato la storia di dei vari Paesi occidentali dell'Europa? Come fate a non capire cosa sta accadendo al partito socialista francese, a quello spagnolo, ai partiti che a vario tipo sono stati legati ai grandi gruppi politici di questi decenni, come i popolari e i socialisti? È possibile che vediamo solo noi che quel sistema politico che ha segnato una grande parte della storia, e non soltanto della Repubblica italiana ma dell'intero continente europeo, si sta drammaticamente sgretolando sotto ai vostri e ai nostri occhi? Come fate a non vedere che sta crollando un intero sistema politico? Quando succede una cosa come questa, davvero bisognerebbe contare fino a tre prima di parlare. In una situazione che ha siffatte caratteristiche, caratteristiche, tali da poter travolgere l'intero sistema politico, io trovo del tutto irresponsabile fare una scelta come questa, nel metodo. Non si cambia la legge elettorale a pochi mesi dal voto.

esterno all'attuale Parlamento, che potrebbe avere tutto il diritto di dire che le regole democratiche non si cambiano a poche settimane dal voto. Addirittura però finanche con la contrarietà di quello che - ci piaccia o meno - è comunque il più grande partito o movimento di opposizione del Paese,

con "Italia. Bene Comune", una coalizione che metteva assieme le forze democratiche e progressiste del Paese: il Partito Democratico e all'epoca Sinistra Ecologia e Libertà.

una lontananza sempre maggiore di quello che fu il nostro alleato cinque anni fa, il Partito Democratico, dal mondo che all'epoca cercammo di rappresentare insieme. Forse - come dice qualcuno è un bene, perché non bastano più gli album di famiglia per creare le coalizioni politiche. Gli album di famiglia non esistono più. Credo che la scelta che avete fatto stasera sia l'epilogo finale di una precisa traiettoria politica. La stagione del renzismo ha chiuso qualunque rapporto di quel partito che un tempo fu nostro alleato con la sinistra italiana, quella con la "s" minuscola, non quella con la "S" maiuscola. Voglio quindi

dare un'altra opportunità ai cittadini di questo Paese e farlo attraverso una piattaforma politica radicalmente alternativa alla vostra, colleghi del Partito Democratico. Sono molto convinto del fatto che, esattamente come è successo qualche mese fa, quando eravate maggioranza in questo Parlamento, ma totale minoranza nel Paese, ancora una volta, da qui a pochi mesi, sarete stati maggioranza qui, ma sarete minoranza fuori.

anche qui al Senato, dopo che questa sciagurata decisione è stata presa alla Camera dei deputati. So che voi state ridendo di noi. Vi ho visti ridere Ma che cosa importa ai disoccupati, ai cassintegrati e ai giovani che non trovano opportunità della fatua battaglia parlamentare delle opposizioni sulle poltrone? Questo è il vostro ragionamento, ma vi sbagliate di grosso. Le donne e gli uomini di questo Paese, i nostri concittadini, sono più intelligenti di come voi li fate e ve l'hanno dimostrato il 4 dicembre Forse non conoscono bene i Regolamenti parlamentari e il galateo istituzionale che voi oggi violentate, ma una cosa l'hanno capita benissimo: quando le poltrone sono le vostre, la fiducia la mettete e il risultato lo portate a casa. Metterete forse la fiducia per punire le imprese che delocalizzano in Polonia o in Romania? No di certo. Metterete forse la fiducia per stabilizzare i ricercatori precari degli enti di ricerca? No di certo. Metterete forse la fiducia per introdurre norme sull'educazione sentimentale e di genere, per combattere quotidiani stupri e femminicidi a opera di nostri concittadini che hanno un concetto malato delle donne? No di certo. Metterete forse la fiducia per assumere i giovani competenti e motivati nelle pubbliche amministrazioni e superare il blocco del *turnover*? No di certo. Metterete forse la fiducia sul No di certo. Metterete forse la fiducia sull'abolizione del *superticket* negli ospedali pubblici? Mettete forse la fiducia per non alzare l'età pensionabile? No di certo. No, colleghi, la questione di fiducia non la mettete mai

Ma vi sbagliate di grosso, perché gli italiani non sono affatto degli stupidi: lo hanno dimostrato il 4 dicembre scorso e lo dimostreranno alle prossime elezioni

mi rivolgo ai cittadini italiani per dire loro cosa produrrà il disegno di legge elettorale in esame, che qualcuno ha rinominato Fascistellum per via dei cinque voti di fiducia con i quali è stato approvato alla Camera dei deputati e sul quale porrete la fiducia anche qui in Senato. certamente dichiarato incostituzionale, così come il Porcellum, l'Italicum e i tanti decreti che avete adottato. Tuttavia, per capire quali saranno gli effetti di questo disegno di legge elettorale dobbiamo ripercorrere un po' quanto accaduto. L'8 settembre 2007, dieci anni fa, in tutte le piazze d'Italia si celebrò il primo V-Day. C'ero io e c'eravamo tutti noi del Movimento 5 Stelle. Chiedevamo il divieto di candidatura in Parlamento per i condannati, in via definitiva e non, per reati per reati non colposi con pene superiori a dieci mesi e venti giorni; il limite di due legislature per i parlamentari; la modifica della legge elettorale attraverso l'introduzione del voto di preferenza. Se queste cose semplici e di buon senso fossero state prese in considerazione dalla politica, noi oggi non saremmo qui. Marzo 2013: il Movimento 5 Stelle entra in Parlamento. Elezione del nuovo Presidente della Repubblica, dopo Giorgio Napolitano: il Movimento 5 Stelle propone e vota Stefano Rodotà e, mentre la piazza qui fuori urlava il suo nome («Rodotà, Rodotà!»), voi, pensando di salvare poltrone e potere, rivotate, come mai era successo prima nella storia, per la seconda volta di seguito lo stesso Presidente della Repubblica, ancora Giorgio Napolitano. Aprile 2013: nasce il Governo tra PD e Forza Italia. Letta e Alfano formano il primo Governo di questa legislatura, il PD inizia la sua crisi. 4 Dicembre 2013: la Corte dichiara incostituzionale il Porcellum, la maggioranza in Parlamento è abusiva. I cittadini e il Movimento 5 Stelle chiedono subito nuove elezioni, che non arriveranno. Successivamente, Napolitano incarica Letta di riformare la Costituzione e nomina un comitato di saggi con la volontà di scardinare la Costituzione attraverso la modifica dell'articolo 138. I partiti conducono una campagna d'odio nei confronti della Costituzione. Ma il Movimento 5 Stelle, nel silenzio totale dei *media*, sale sul tetto di Montecitorio e salva la Costituzione. Febbraio 2014: Napolitano caccia via Letta per non essere riuscito a smontare la Costituzione. Poi prende Renzi e la Boschi e gli affida lo stesso compito: andate e distruggete la Costituzione. Aprile 2014: loro, da bravi servi di corte, procedono, iniziano dalle Province: fanno credere di averle abolite e invece cancellano solo il voto dei cittadini. Sempre nell'aprile 2014 Renzi e Boschi depositano la riforma costituzionale, ma gli andrà male, molto male. Maggio 2015: con i voti di fiducia e grazie al patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi, viene approvato l'Italicum. Il PD continua a perdere pezzi, elettori, faccia, tutto. 4 Dicembre 2016: gli italiani, con il 60 per cento dei voti contrari, disintegrano la riforma sovversiva della Costituzione italiana che portava la firma del PD, si liberano di Renzi e della Boschi e mandano un messaggio chiaro: non vi vogliamo più, andatevene. Il 10 dicembre 2016, dopo essere stati ricevuti dal Presidente della Repubblica per le consultazioni dei Gruppi parlamentari, al termine dell'incontro, i capigruppo del Movimento 5 Stelle Luigi Gaetti e Giulia Grillo ribadivano la nostra assoluta contrarietà al conferimento di un nuovo incarico di Governo. Testualmente «In attesa che la Consulta si esprima sulla legge elettorale, il Governo dimissionario deve limitarsi ad essere mero strumento regolamentare al servizio del Parlamento e soprattutto della Corte costituzionale. Qualsiasi altra soluzione sarà un tradimento della volontà popolare. Non si può abusare oltre ogni misura della pazienza dei cittadini. La loro volontà va rispettata, non violata». Lo stesso giorno, al termine delle consultazioni, il presidente della Repubblica Mattarella dirà: «In questi incontri è emersa, come prioritaria, un'esigenza generale di armonizzazione delle due leggi per l'elezione della Camera e del Senato, condizione questa indispensabile per procedere allo svolgimento di elezioni». L'11 dicembre 2016 Paolo Gentiloni Silveri riceve l'incarico dal presidente Mattarella, il 12 dicembre rinomina gli stessi Ministri del Governo Renzi, prendendo in giro gli italiani. Gennaio 2017: la Consulta dichiara incostituzionale l'Italicum, dichiara incostituzionale il ballottaggio e la possibilità per i capilista bloccati di scegliersi il collegio di elezione. In pochi minuti ho elencato solo In pochi minuti ho elencato solo alcuni dei danni che avete combinato in questi cinque anni e non ho parlato nemmeno di *jobs act*, buona scuola, sfascia Italia. Questo breve resoconto per dimostrare quanto siete stati irresponsabili. Non saranno i voti di fiducia qui dentro a salvarvi dal giudizio dei cittadini, perché la vera fiducia che serve è lì fuori, nelle piazze, tra la gente, e voi non ce l'avete. Questa legge elettorale infame, che priva i cittadini della possibilità di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento, avrà due effetti a breve tempo. Il primo effetto lo vedrete il 5 novembre prossimo in Sicilia, dove i cittadini,

sia per l'oggetto, la legge elettorale, sia per il clima conflittuale che, ancora una volta, caratterizza un passaggio cruciale della vita parlamentare. Abbiamo ormai da tempo lasciato alle spalle il criterio guida della sistematicità e della coerenza tra forma di Governo, sistema parlamentare e legge elettorale. Gli approcci proporzionali avevano una volta una propria linearità; così gli approcci elettorali maggioritari. Via via, nel mondo, abbiamo conosciuto correttivi e sistemi misti. In Italia siamo arrivati in ritardo. I sistemi elettorali dei Paesi avanzati questi nodi li hanno saputi sciogliere dopo la Seconda guerra mondiale e oggi hanno più storia ed energia democratica per affrontare le tremende sfide delle crisi sociali ed economiche, il risorgere devastante dei populismi, il dilagare delle tante ingiustizie presenti nella globalizzazione senza regole. Il cammino della Seconda Repubblica è stato, anche da questo punto di vista, tormentato. Eravamo partiti abbastanza bene con il Mattarellum. Poi, via via, ci siamo persi, sino ad arrivare a votare, dal 2006, con il cosiddetto Porcellum. Insomma, la crisi della politica è entrata dentro, sino al midollo del sistema democratico. Ha travolto definitivamente il sistema antico e oggi tanto rimpianto del partito Noi, protagonista della Prima Repubblica, e ci ha lasciato in balia del fallimentare e distruttivo partito Io dell'attuale Seconda Repubblica. Così oggi abbiamo una seria difficoltà a venirne fuori. È vero nel Rosatellum si continua a rinunciare ad un punto qualificante del principio di rappresentanza: la probabile e realistica possibilità, il giorno dopo le elezioni, di avere una chiara maggioranza intorno cui dotare il Paese di un Governo stabile. Questa onesta e semmai scontata critica non mi induce a difendere l'attuale legge elettorale: niente di tutto ciò. Difendere o accettare passivamente il Porcellum-Consultellum in vigore è il vero punto debole di chi oggi si oppone, anche con veemenza, al Rosatellum. Non penso che sia una buona scelta andare a votare con una legge non votata dal Parlamento, visto che il Consultellum è il prodotto dell'inevitabile intervento della Corte costituzionale. Capisco che di questi tempi reclamare uno dei fondamenti della democrazia, che prevede che sia il Parlamento a votare la legge elettorale, non è un valore da apprezzare. di là, però, del valore, anche sul piano più terra terra della efficacia minima da richiedere a una legge elettorale, con il Consultellum dovremmo andare a votare con una legge del tutto asimmetrica tra Camera e Senato. Una diversità astrusa e incomprensibile, che rischia di essere rovinosa e di dare un colpo mortale alla vita democratica del nostro Paese, senza in cambio dare nessun beneficio, come, ad esempio, dare la possibilità di formare un Governo in modo trasparente e con coalizioni coerenti. Nella legge che ci apprestiamo a varare, l'asimmetria tra Camera e Senato viene positivamente superata: non è cosa da poco. Collegi uninominali sia alla Camera che al Senato, con grandezze naturalmente diverse, e collegi plurinominali, altrettanto coerenti, per le due Camere. Un altro aspetto positivo del Rosatellum non va sottovalutato: viene recuperato, seppur parzialmente, il meccanismo coalizionale, incentivato dalla previsione di collegi uninominali, con un certo peso maggioritario che ne scaturisce. Rimane un punto non risolto. Si lascia, nella parte proporzionale, la lista bloccata: un errore, un limite che non fa bene alla politica e alla necessità di selezionare una più radicata e autorevole classe dirigente e parlamentare. Cari colleghi, siamo ancora in una incancrenita fase di transizione. La Terza Repubblica non decolla. Nella prossima legislatura, il Parlamento dovrà lavorare al Paese un assetto istituzionale capace di coniugare decisione democratica e partecipazione democratica. Due valori regolativi che debbono vivere insieme e orientare le scelte di fondo di una solida e matura terza fase della nostra Repubblica. Anche il clima politico dovrà essere diverso: più cooperazione e più responsabilità. In molti di noi parlamentari della maggioranza rimane una riserva sulla scelta di porre la fiducia, è innegabile, e anche la volontà di votare questa legge elettorale è tutta giocata sulla riduzione del danno. È già un risultato che va comunque apprezzato e condiviso.

abbiamo imparato che non ci sono *leader* salvifici che possano risolvere da soli i problemi di tanti e che l'informazione di giornaloni e televisioni sono spudoratamente asservite e lì vi troviamo e vi ascoltiamo il contrario di ciò che è vero. La chiave del cambiamento sta nella partecipazione, una consapevolezza ormai chiara, anche sottolineata dal voto referendario che ha rispedito al mittente la "deforma costituzionale "ispirata al modello dell'uomo solo al comando. È maturata nel Paese la consapevolezza che esiste un'alternativa possibile a quelle politiche stravolgi liberiste - altro che neoliberiste! - di precarizzazione del lavoro, mercificazione dei diritti e cancellazione dello Stato sociale, che, tra l'altro, hanno attraversato in questi anni gli ultimi Governi. C'è un popolo vastissimo pronto a sostenere una forza politica come la nostra che se ne faccia interprete. Abbiamo segnato una netta rottura con il passato: ridare protagonismo alla partecipazione dei cittadini, rivendicare senza compromessi i diritti che ci sono stati tolti per costruire una società più giusta, inclusiva e realmente fondata sul riconoscimento dei talenti e sulla solidarietà sociale, in grado di contrastare le riforme dettate dalle rapaci *lobby* capitalistiche senza scrupoli e da Governi deboli e consenzienti e forze politiche autoreferenziali. La nostra forza politica è l'unica capace di invertire la rotta a questo modello di sviluppo, fondato sulla cancellazione dei diritti e sullo sfruttamento cieco e dissennato dell'ambiente, del territorio, delle risorse artistiche e culturali del nostro Paese. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che rappresenta i diritti e le ragioni del lavoro, delle giovani generazioni lasciate da voi senza futuro, della vecchia classe media che non esiste più, per colpa vostra. In questi anni, da opposizione finalmente benvenuta opposizione, anche in Italia - abbiamo lottato per i diritti e abbiamo fatto proposte concrete e alternative, con coraggio e senza compromessi. Siamo ad una nuova legge truffa? Sì, siamo ad una nuova legge truffa, anzi criminale. Questa legge è palesemente una violazione della libertà di voto, come ha detto anche Paolo Mieli, persona che notoriamente non sta dalla nostra parte, anzi. Questa legge è pensata per penalizzare la volontà popolare e per di più è varata a pochi mesi dalle elezioni, con chiaro intento di truccare il risultato e non essere bacchettati da chi potrebbe potrebbe farlo, cioè la Corte costituzionale, che non ne avrà il tempo. È il vergognoso prodotto di una maggioranza eletta con una legge incostituzionale, il Porcellum, che avendo fallito con l'Italicum adesso ritorna con l'obiettivo di blindarsi sempre di più in Parlamento con questa nuova legge elettorale, in modo poi da governare, destra e sinistra, come hanno sempre fatto, con le famose ammucchiate, nascoste però da parole per reiterare le sciagurate politiche neoliberiste, per continuare a spremere e disprezzare ancora di più i lavoratori e i piccoli e i piccoli e medi imprenditori. Lo scopo non è dare una legge elettorale più giusta al Paese - il Consultellum con soglie equiparate tra Camera e Senato sarebbe stato più che sufficiente - ma favorire un Governo di larghe intese PD e destre; impedire agli italiani di scegliere candidati ed eletti; mortificare l'unico partito di opposizione, cioè il Movimento 5 Stelle. Ci manca solo di vedere Berlusconi alla Presidenza della Repubblica e il quadro sarà completo. Il dramma è che, nella preoccupazione di mantenere ben saldo il potere nelle loro mani, hanno ulteriormente minato la fiducia dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni, questi traditori e corrotti. Si sente molto parlare della crisi della sinistra; i fatti dimostrano che non è la sinistra ad aver perso gli argomenti, anzi, anzi, ce ne sono fin troppi. Il fatto grave è che quelli (partiti, sindacati, società civile) che dovrebbero rappresentarla, portando avanti le istanze dei poveri e degli sfruttati, si sono si sono invece arresi e consegnati con armi e bagagli alle *lobby* finanziarie. Punto. Fine. Si sono fatti una legge elettorale che li avvantaggia. Ma io confido molto nel sentimento partigiano, e poi non hanno messo in conto che non tutti i cittadini sono non tutti i cittadini sono inerti. Gli italiani non sopporterebbero nessuna riedizione di film già visti. La chiave del cambiamento sta nella partecipazione, Presidente. Confido nel senso di responsabilità di tutti. La posta in gioco è molto alta, troppo alta. Non abbiamo paura di sparire,

sono tempi difficili, con ogni evidenza. questo nuovo disegno di legge elettorale come la prosecuzione di un disegno, che non è iniziato in questa legislatura ma che in questa legislatura sembra voler raggiungere il compimento, cioè la sterilizzazione del Parlamento come controllore dell'operato del Governo. A mio avviso, nel dettato della nostra Costituzione è il Parlamento il *dominus* di tutto l'ordinamento costituzionale. La nostra è una Costituzione che presenta uno sbilanciamento forte a favore del Parlamento: il Parlamento influisce sul controllo del potere giudiziario; il Parlamento fa le leggi; il Parlamento controlla l'operato dell'Esecutivo e dal Parlamento viene eletto il garante della Costituzione, nella figura del Presidente della Repubblica. Questo disegno, che era volutamente tirannofobo dopo il Ventennio fascista, aveva però una falla

lo era perché era la fotografia del popolo, del corpo elettorale; lo era perché era eletto o immaginato come eletto con il sistema proporzionale e lì tutto aveva un senso: aveva un senso il *quorum* per modificare la Costituzione, aveva un senso il *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, perché quel Parlamento era la fotografia del popolo. Da quando però questa Repubblica ha cominciato a camminare e a procedere,

truffa e nel 1963 con la modifica dell'articolo 60. Ricordo che, inizialmente, il Senato aveva una durata di sei anni, diversa da quella della Camera; figurarsi se si poneva il problema di avere lo stesso sistema tra Camera e Senato. Perché? Perché quel Parlamento avrebbe dovuto occuparsi di fare delle leggi, di fare un'analisi approfondita, prima di quelli leggi, di trovare una sintesi per esse e di esprimere un Governo che che in qualche modo si mettesse in una posizione servente rispetto al Parlamento. Invece, si è teso sempre più a semplificare; lo si è provato a fare con la riforma fatta dal centrodestra e poi bocciata dall'elettorato, si è continuato a farlo con i tentativi della bicamerale, lo si è continuato a fare ad inizio di questa legislatura e, grazie a Dio, il popolo è stato più lungimirante dei suoi rappresentanti o quantomeno della sua rappresentanza passata dalla legge maggioritaria. Il timore che, ricordo, segnalammo al popolo e al corpo elettorale in occasione del *referendum* costituzionale, era quello del combinato disposto, cioè la sterilizzazione del Senato, che era impossibile assoggettare ad un premio di maggioranza nazionale e il maggioritario alla Camera. Con il maggioritario infatti il Parlamento diventa una sorta di cassa armonica del Governo, una sorta di *airbag* del Governo: il Governo decide e il Parlamento si assume la responsabilità, in pratica, abbiamo un Supergoverno e un Parlamento che ratifica. Questo tipo di impostazione è quella che si otterrà se questa legge verrà approvata; avremo due Camere che avranno una rappresentanza che non sarà proporzionale, ma falsata, che non che non ospiterà rappresentanti dei cittadini voluti in modo diretto, perché con mille ingegnerie ingegnerie si farà in modo che non sia così. Sappiamo infatti che un terzo verranno eletti con l'uninominale, due terzi verranno eletti a strascico, come qualche collega ha detto poc'anzi. Il rapporto tra rappresentato e rappresentanti si allenta. È questo quello che serve? Bisogna capire a chi serve. Il popolo italiano ha rappresentato in ogni modo legittimo possibile il sentimento di disagio per il distacco dai propri rappresentanti, mentre i potentati economici e una certa classe politica, qui rappresentata purtroppo in modo maggioritario, in questo momento, invece chiede una sorta di scioglimento dai lacci e lacciuoli della rappresentanza. È una scelta lungimirante? A mio avviso no. no. Laddove le istanze popolari non vengano recepite dalle Camere, dove dovrebbero essere rappresentate, esse crescono

grave per tutti, anche perché i rivolgimenti violenti si rivolgono anche contro coloro che li hanno fatti partire.

Colleghi, stiamo creando i presupposti per quelle che Cicerone chiamavo *res e francamente la cosa mi impensierisce e mi preoccupa e non capisco come non preoccupi gli altri. Non capisco come non preoccupi la maggioranza dei colleghi, che hanno tutti, generalmente, più esperienza di me in questo ambito. Pertanto vorrei associarmi a chi, prima di me, ha chiesto a quei colleghi della maggioranza, che sono più sensibili a questi temi, di riconsiderare la propria posizione, perché la prima obbedienza la dobbiamo, prima ancora che ai partiti che ci hanno fatto eleggere, alle istituzioni repubblicane

è una dichiarazione di guerra alla sovranità popolare, è una sfida dei partiti a tutti i cittadini che amano la democrazia. Come si fa a definire legge un testo che in più parti è chiaramente incostituzionale? Come si fa a definire elettorale qualcosa che, di fatto, impedisce agli elettori di scegliere i propri rappresentanti alla Camera dei deputati Durante le audizioni si sono palesati almeno sei profili di incostituzionalità. È mai possibile che gli italiani debbano votare con una legge tanto complicata da richiedere lezioni di diritto per essere compresa? Voi state preparando un disastro democratico, perché molte persone andranno a votare senza avere idea di come funziona davvero la legge elettorale e senza capire dove andranno a finire i loro voti. Al posto di una scheda elettorale, gli italiani si ritroveranno con un contratto incomprensibile, con tanto di bugiardino: qualcosa che ricorda tanto i complicatissimi contratti con cui le banche - a voi care - hanno truffato i risparmiatori, convincendoli ad

Quando qualcosa è troppo complicato per essere capito immediatamente, allora potete stare sicuri che sotto c'è la fregatura. I partiti si illudono che gli italiani non mangino la foglia, ma si sbagliano di grosso, come si sono sbagliati lo scorso 4 dicembre, quando 20 milioni di cittadini hanno sventato il tentato furto, con scasso, della Costituzione. Signor Presidente, voglio fare almeno un paio di esempi chiari, per dare un'idea di quanto siano subdoli i vostri stratagemmi per rimanere attaccati alle poltrone: se un elettore di Fratelli d'Italia metterà la croce sul nome di Giorgia Meloni, il suo voto andrà sì alla Meloni, ma sarà anche spalmato maggiormente su Forza Italia e Lega, che incasseranno molti più voti di quelli realmente espressi dagli elettori.

Faccio un secondo esempio: un signore che, suo malgrado, non può più sedere in quest'Aula, si è inventato un movimento animalista; quando gli elettori metteranno la croce sul movimento animalista, perché comprensibilmente preferiscono cani e gatti a questa classe politica con la soglia del 3 per cento, inconsapevolmente, daranno il loro voto, di fatto, a Forza Italia e Lega. *Idem* per la coalizione di centrosinistra, se centrosinistra si può chiamare. Un meccanismo ideato per spazzolare i voti degli elettori che mai e poi mai metterebbero la croce sul PD o su Forza Italia, ma che potrebbero metterla su liste civetta come un sedicente partito dei precari o un movimento dei pensionati. Avete capito che gli italiani non vi sopportano più. Avete capito che non vedono l'ora di andare a votare per mandarvi a casa, avete avuto paura e avete escogitato una legge elettorale, anzi, chiamiamolo col suo nome, un imbroglio, attraverso il quale vince chi perde. Una truffa diabolica per dirottare il voto degli elettori dove più vi conviene. In cinque minuti è impossibile spiegare nel dettaglio tutte le storture del Rosatellum, ma almeno un'altra cosa reputo sia obbligatorio dirla. Vi siete vantati del fatto che il Rosatellum recupera il rapporto fra eletto e territorio, che gli elettori, grazie alle liste corte di candidati, possono conoscere i nomi a cui andrà il loro voto. Falso! Doppiamente falso! Intanto, nei listini proporzionali sono previste le pluricandidature, quindi lo stesso candidato può essere infilato contemporaneamente a Bergamo e a Caserta. Altro che legame con il territorio! Seconda cosa, i listini corti sono solo una finzione, perché in realtà i listini sono ancora più lunghi lunghi di quelli previsti dal Porcellum. Per un effetto di slittamento, il mio voto può essere usato non per assegnare il seggio a uno dei nomi che ho trovato nella mia lista, ma per assegnarlo a uno dei nomi presenti nelle liste di tutta Italia, visto che viene ripartito in modo proporzionale a livello nazionale. Quindi, per quanto l'elettore ne sa, il suo voto, dato a una lista di persone di suo gradimento, può essere travasato e utilizzato per dare il seggio a un impresentabile candidato a centinaia di chilometri di distanza,